come ogni anno il decreto chiamato milleproroghe affronta temi non arrivati a soluzione e presenta ovviamente soluzioni per porvi rimedio. Vorrei soffermarmi sulle tante e diverse tematiche affrontate dal decreto e dalle modifiche inserite in sede parlamentare che riguardano la mia Regione e i temi che ho seguito, alcune specifiche e dedicate, altre che coinvolgono specificità nella mia Regione, la Sicilia. Vorrei cominciare dal nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa. La norma contenuta nel decreto consente la realizzazione del polo ospedaliero, prorogando da due a tre anni il termine per la sua realizzazione. Ugualmente, viene prorogata di un ulteriore anno anche la figura del commissario straordinario, che è stato appunto nominato allo scopo di realizzare il polo ospedaliero. una norma attesa, posto che lo scorso 25 gennaio è stato pubblicato l'avviso d'indagine di mercato per la definizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria, finalizzato alla progettazione definitiva per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. L'auspicio è quindi che ora si vada avanti spediti e che si possano dotare i nostri territori di un moderno presidio ospedaliero a tutela della salute dei cittadini e di tutto il comprensorio. Vi sono poi norme che riguardano Lampedusa e Linosa, che fissano al 30 giugno e al 30 novembre il termine dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scaduti fino al dicembre 2020. I versamenti possono essere rateizzati e pagati senza interessi, dando in questo modo una boccata di ossigeno a molti contribuenti di quei territori così colpiti. A favore di Linosa e Lampedusa vengono anche stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Viene prevista poi la possibilità di distribuire fino al 31 marzo alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina il contributo di 40 milioni previsto dall'ultima legge di bilancio, quella approvata a dicembre. è poi la norma che prevede il passaggio delle competenze di commissario della baraccopoli di Messina al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in sostituzione del prefetto di Messina. Questo è un tema su cui Forza Italia ha fatto tanto sin dalla passata legislatura, battendosi affinché si smantellasse quella baraccopoli, rimasta in piedi troppi anni. Dopo tanti anni, è arrivato il momento di portare a termine la riqualificazione urbana dell'area su cui appunto si trovavano le baracche, dove molta gente ha vissuto a lungo, quasi come se fosse una cosa normale. una tematica che riguarda ancora migliaia di persone, cui bisogna dare la dignità di vivere in una casa normale. Speriamo questo accada entro il prossimo anno. Apprezziamo in particolare anche la disposizione che consente agli studenti universitari fuori sede, ai disabili gravi, ai lavoratori fuori sede con un reddito basso e alle persone che dalla Sicilia migrano per motivi di salute e di lavoro di accedere a un contributo per i biglietti aerei per i voli da e per Catania e Palermo. È un'attenzione volta a garantire la continuità territoriale per soggetti specifici, che non possono rimanere isolati per il solo fatto di vivere in un'isola. È inoltre prevista una proroga che prevede che la riorganizzazione del sistema delle camere di commercio della Sicilia possa avvenire entro la fine dell'anno. sono poi le norme che riguardano lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Le disposizioni consentono di impiegare risorse correnti non utilizzate, per avvalersi di strutture private accreditate, e di derogare ai regimi tariffari ordinari. La Sicilia è purtroppo tra le Regioni sottoposte al Piano di rientro da disavanzo sanitario, ma la salute dei cittadini viene e deve venire prima di tutto. Questa disposizione consente quindi di gestire al meglio le tante richieste di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini ed è certamente una norma attesa e benvenuta, peraltro, in un contesto che tiene a mente che il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve garantire ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità.

nazionale, che vale 50 milioni di euro, 10 milioni per ciascuno degli anni che vanno dal 2023 al 2027, a sostegno di un piano prontamente predisposto dal ministro Schillaci e immediatamente finanziato dal Parlamento, che ha dato il suo consenso pressoché unanime. piano potrà aiutare migliaia di pazienti ad avere un sistema di cure più omogeneo sul territorio nazionale, incluse le Regioni del Sud, che storicamente scontano ritardi e una migrazione legata a motivi di salute verso le Regioni più organizzate ed efficienti. Sempre in tema di salute, va bene la proroga del Patto per la salute 2019-2021, fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Insomma, vanno colmati alcuni ritardi e certamente per farlo occorre il tempo opportuno. Sono felice per l'approvazione dell'emendamento che proroga i termini per la stabilizzazione del personale sanitario proprio per rafforzare il sistema sanitario, fronteggiando la grave carenza di personale.

e poi delle Commissioni riunite del Senato, che ci hanno visti impegnati in diverse sedute e che hanno registrato l'accoglimento di molte nostre proposte emendative. Insieme siamo riusciti a individuare una serie di tematiche cui dare una soluzione e devo dire che l'ascolto del Governo e dei relatori è stato molto attento e pronto a recepire le proposte nell'interesse dei cittadini e delle nostre comunità.

speravamo davvero che, in occasione della conversione del decreto-legge milleproroghe, il Governo cogliesse l'opportunità di rimediare alla legge di bilancio, che ha evidenziato chiaramente la totale la totale inadeguatezza dell'Esecutivo a far fronte, con responsabilità e determinazione, alle emergenze economiche e sociali del nostro Paese. Colleghi, in questo decreto-legge troviamo anche alcune misure apprezzabili, già introdotte e difese dal MoVimento 5 Stelle: mi riferisco alla proroga del termine per accedere ai mutui agevolati per la prima casa per le giovani coppie; alla proroga del termine per consentire alle imprese di usufruire dei crediti d'imposta relativi a transizione 4.0; alla proroga dell'utilizzo delle ricette sanitarie elettroniche e al rinnovo dei medici specializzandi per sopperire alla carenza di personale negli ospedali. sicuramente meritoria anche la proroga dello *smart working* per i lavoratori fragili, fortemente voluta da tutte le forze politiche in Commissione.

Sarebbero tanti, direi troppi, gli esempi da citare di tutti i mancati provvedimenti che impattano sulle fasce più deboli del nostro Paese. A cosa mi riferisco, colleghi? Penso alla mancata proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, che di fatto con il caro benzina va a incidere sull'aumento dei costi per i trasportatori

Penso alla mancata proroga del termine del regime transitorio del reddito di cittadinanza, che ad agosto verrà tolto ai cosiddetti occupabili, senza che nulla sia ancora stato fatto per i fantomatici corsi di formazione che avrebbero dovuto che avrebbero dovuto garantire ai circa 600.000 percettori occupabili di trovare finalmente un posto di lavoro. Tra tutte le occasioni perdute, una delle più macroscopiche e - aggiungo è la mancata proroga che avrebbe potuto fare la differenza per 40.000 imprese a rischio di fallimento a causa di tutti gli sciagurati interventi sul superbonus al 110 per cento. *(Applausi)*. Presidente, questo è un dato drammatico. Infatti, sulla necessità di un intervento per sbloccare i crediti Giorgia Meloni ha fatto campagna elettorale. Fratelli d'Italia è sceso in piazza, è andato alle manifestazioni per l'edilizia, salvo poi tradire chi l'aveva votato per questo. una delle tante promesse non mantenute dalla maggioranza e dal Governo. Il Governo si giustifica dicendo che non ci sono le risorse per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Peccato però che i soldi si trovano, quando si devono fare contenti gli amici di Lotito, per esempio con le società di calcio di serie A. *(Applausi)*. Oppure le risorse non si vogliono trovare: guai a parlare della tassazione degli extraprofitti, che avrebbe portato dai 10 ai 12 miliardi nelle casse dello Stato per la collettività, per tutti i nostri concittadini. un dato drammatico, perché il balletto in Commissione sull'emendamento prima presentato da Fratelli d'Italia sulla proroga del superbonus per le villette unifamiliari, poi ritirato su richiesta del Governo, la dice lunga su chi tiene i cordoni della borsa e decide realmente in seno all'Esecutivo. *(Applausi)*. È drammatico perché la direttiva europea sulle case *green*, prima che un impegno, rappresenta per l'Italia un'occasione storica di sviluppo nella direzione della transizione ecologica e di impulso alla creazione di posti di lavoro; tratta di un impegno che avrebbe creato posti di lavoro e che avrebbe portato un aumento del PIL; un impegno che il nostro Paese avrebbe assolto in scioltezza grazie al superbonus al 110 per cento,

direttiva. È il caso di ricordare a chi ci sta ascoltando che tale direttiva è stata votata ed ha avuto il via libera del ministro dell'energia Pichetto Fratin, che ha approvato il testo insieme ai suoi omologhi in Europa. C'è di più, signor perché oltre che un'occasione persa, quella del superbonus è l'ennesima giravolta e prova di incoerenza della maggioranza e di Giorgia Meloni, una maggioranza che in campagna elettorale e a giorni alterni al Governo - e l'abbiamo sentito anche ieri dai banchi della maggioranza venti che sbloccare i crediti incagliati delle imprese è una priorità. Allora cosa fa il Governo di Giorgia Meloni? Quando ha l'occasione di mantenere una promessa, ingrana la retromarcia e volta le spalle a imprese e lavoratori. Lo sanno bene le imprese, che già stanno facendo partire le prime lettere di licenziamento dei lavoratori assunti grazie al superbonus; lo sanno bene le famiglie, che si stanno indebitando per poter vedere l'ultimazione dei lavori nelle proprie abitazioni. l'ufficio statistico dell'Unione europea, ieri in Commissione finanze ha chiaramente detto che sono stati i ripetuti interventi che hanno cambiato la norma ad avere incagliato i crediti: insomma, il superbonus era stato scritto bene, sono stati gli interventi successivi che l'hanno rovinato e l'hanno reso inefficiente. *(Applausi)*. Eurostat ha precisato che la cedibilità non impatta sul debito, ma solo sul *deficit*, e ha una ricaduta positiva sull'economia,

i fatti inoppugnabili portati ieri in Commissione finanze da Eurostat inchiodano Meloni e Giorgetti alle loro responsabilità per l'ennesima promessa non mantenuta. Quindi, in che modo il Governo pensa di creare sviluppo? Mettendo a rischio i 900.000 nuovi posti di lavoro creati dal superbonus? Mettendo in ginocchio le imprese e l'indotto del settore edilizio? In che modo il Governo pensa di condurre il Paese verso il futuro di una vera transizione ecologica? Facendo un'inversione a U rispetto al percorso tracciato e sottoscritto in Europa? Ma quale coraggio, quale visione del futuro! Questo è un Esecutivo saldamente ancorato al passato di una politica di austerità, che privilegia pochi a discapito di tutti gli altri cittadini *(Applausi)* e che continua a generare differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, tra Regioni di serie A e Regioni di serie B. Mi avvio alla conclusione, Presidente: vi ricordate la nave nel mare in tempesta evocata da Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia? Ebbene, ad oggi, sul ponte di comando di questa nave in tempesta si sente riecheggiare un solo ordine: indietro tutta!

al dibattito. Questo ci era stato chiesto in particolar modo dai colleghi della minoranza, che probabilmente non hanno potuto, neanche quando erano della maggioranza, scendere nell'agone politico e valorizzare il dibattito politico neanche quando erano al Governo, con i loro rappresentanti seduti sugli scranni più importanti. hanno chiesto di far tornare il Parlamento protagonista: questo è accaduto con un'audizione

al Governo e al ministro Ciriani per un lavoro incredibile di triangolazione nel merito, che abbiamo portato avanti per riuscire a far tornare

della scuola si è detto, così come degli enti locali, per quanto riguarda i Comuni in disavanzo, e delle strutture turistiche, sia per l'antincendio, sia per il sostegno alle stesse. L'ultima sera, quella che precede l'approvazione finale, in Commissione abbiamo avuto un gesto fortissimo, che porta la firma del presidente Meloni, ma che è stato fortemente voluto dal presidente Guidi

Il presidente Meloni ha voluto, nell'ultima notte, che si reperissero 16 milioni di euro per prorogare lo *smart working* per i fragili. Questo è stato ottenuto e credo sia stata una vittoria di civiltà, di tutto il Parlamento e non soltanto della maggioranza.

alla proroga di un anno dei cosiddetti tribunali minori, nella misura in cui tanto il ministro Nordio, quanto il sottosegretario Delmastro Delle Vedove hanno riconosciuto l'importanza dei presidi di legalità e dell'erogazione di servizi così importanti

al sottosegretario Gemmato, per completare la filiera con il ministro Schillaci. Finalmente la sanità non è più ideologizzata,

proprio perché rivolta a un aspetto e a uno spaccato della società che sono coinvolti a 360 gradi nella tematica della patologia oncologica poi ne pagano le conseguenze, non soltanto con riferimento ai diretti interessati, ma anche alle famiglie e a tutti coloro che vengono in vario modo interessati da una patologia, che è invalidante per se stessi e per chi li circonda. Accanto al piano oncologico nazionale, cito le misure sulle liste d'attesa, che sono importanti per la prevenzione e per la diagnosi precoce e per evitare che

poi attenzione nei confronti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui c'è grande carenza nei territori, in particolar modo nelle aree montane, nelle aree interne e nei piccoli borghi. Da la doppia misura per consentire ai giovani medici di sostituire e di prendere incarichi provvisori, per quanto riguarda i medici di medicina generale, e agli specializzandi dei primi anni, per quanto riguarda i pediatri di libera scelta. Penso altresì alla possibilità di andare in pensione a settantadue anni per gli stessi medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Non abbiamo dimenticato

spesso in maniera inappropriata parlano di luna di miele. Beh, ci sono amori e innamoramenti che non hanno fine: con queste premesse, l'amore nei confronti di Giorgia Meloni, del Governo Meloni e del centrodestra sta andando avanti

Prendiamo atto che non è stato possibile soddisfare tutte le attese,

Nel dibattito sono stati sottolineati gli importanti risultati conseguiti in Commissione con l'approvazione di tantissimi emendamenti; altri, che pure avremmo voluto approvare, non è stato possibile approvarli, perché purtroppo c'è un tema di risorse. Checché se ne dica, bisogna mantenere in ordine

fino in fondo quel senso di responsabilità che magari altri non hanno esercitato quando c'era anche maggior margine rispetto a oggi. Tutto sommato, quindi, il bilancio è molto positivo; l'auspicio è che il confronto prosegua in questo modo anche nell'esame e nella votazione degli emendamenti, perché comunque nel disegno di legge di conversione, oltre che nel decreto-legge, ci sono importantissime misure che hanno urgenza di essere adottate. Ricordo che entro il 27 febbraio anche la Camera dovrà approvare il testo che uscirà dal Senato e mi preme sottolineare, come hanno fatto molti nel corso del dibattito, che che particolare attenzione è stata rivolta, nel corso dei nostri lavori, proprio alle categorie più fragili e più in difficoltà, che ancora faticano a uscire dalla crisi economica dovuta alla sinergia alla sinergia negativa di pandemia e crisi ucraina. In conclusione, ringrazio tutti e spero che si possa concludere al più presto con tale spirito la votazione su questo importante provvedimento.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4-*ter*.0.305 (limitatamente al comma 2),

parere del Governo

prevede semplicemente la proroga di sei mesi - fino al 30 giugno 2023 - del termine ultimo, attualmente previsto per il 31 dicembre 2022, per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti riferite alle risorse assegnate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione rispetto alla programmazione 2014-2020. In tal modo, verrebbero salvaguardati numerosi finanziamenti destinati a interventi strategici pronti a essere messi a gara, che con l'attuale

parere del Governo

dell'emendamento 3.301, che riprende i testi degli emendamenti 11.51, 3.72 e 11.48, presentati in Commissione dalla maggioranza. Immagino che, essendo appunto testi presentati dalla maggioranza che noi abbiamo ripreso per l'Assemblea, avranno ovviamente il parere favorevole della maggioranza, che non voterà contro se stessa.

tutti i colleghi che hanno lavorato con me in Commissione ed il Governo per aver capito che era necessario impegnarsi affinché si arrivasse alla proroga dei termini della stabilizzazione per il personale sanitario

Sono emendamenti a costo zero, perché le stabilizzazioni vengono fatte nell'ambito delle risorse a disposizione degli enti,

per gli operatori sanitari, per gli amministrativi e non per i ricercatori. Sappiamo anche quanto i ricercatori degli IRCCS abbiano dato un contributo fondamentale

tempo al Governo di rivalutare questo *vulnus* e questa incongruenza, perché davvero sono rimasti fuori solo i ricercatori. Speriamo che il parere sia favorevole.

Noi intendiamo con questo emendamento estendere e rendere definitiva l'adozione della ricetta dematerializzata.

ad un'opportunità che ha mostrato tutto il suo valore. Perciò è una richiesta di proroga che renda strutturale questa misura.

Presidente, in Commissione tutti abbiamo auspicato che questa norma possa essere stabilizzata e diventare definitiva. Quindi è un auspicio unanime di tutta la Commissione. Tuttavia la Commissione ha dovuto prendere atto che stiamo parlando di un provvedimento che si intitola "proroga termini". Dunque non si può, in questa sede, perché sarebbe inammissibile, votare l'emendamento come lo propone la senatrice Zampa. Tutti ci siamo augurati che, nel primo provvedimento utile in cui si potrà fare, ciò che oggi la senatrice auspica possa avvenire. Purtroppo non può avvenire in questa sede e sottolineo la parola

in parte ripercorre quanto ha detto la senatrice Castellone. Si tratta di una aggiunta all'emendamento che è stata approvato, con riformulazione, all'unanimità e specifica che, oltre alla possibilità di estendere i termini per la stabilizzazione del personale «sanitario, socio-sanitario e amministrativo», si fa riferimento anche ai profili di «assistente informatico e collaboratore tecnico professionale». Nella precedente formulazione avevamo scritto più genericamente un riferimento ai tecnici e l'obiezione che veniva dal parere contrario del Governo, che ha poi riformulato, era dovuta alla genericità del termine «tecnico». Qui lo specifichiamo e, come ho detto ieri in sede di discussione, è importante ricordare quanto queste figure siano state importanti nel periodo del Covid-19. Quindi faccio riferimento a quanto è stato discusso in Commissione bilancio e al il parere del relatore, conforme a quello del Governo, faceva riferimento alla necessità di una formulazione per invarianza di spesa. Essendo un'estensione di termini per la stabilizzazione, forse questa può essere una possibile riformulazione, se

era sbagliato, ma anche la formulazione corretta, a nostro avviso, deve seguire quell'*iter* che avevamo preventivato in Commissione, che è quello delineato dal presidente Balboni, vale a dire, l'impegno di tutta la Commissione affinché questa questa norma diventi strutturale e non ci sia più bisogno di fare proroghe. Spero che questo impegno che abbiamo preso in Commissione venga rispettato dal Governo e che quanto prima questa semplificazione, che abbiamo introdotto durante la pandemia, per la vita dei cittadini, che finalmente non devono recarsi dal medico di medicina generale per ritirare la prescrizione e che possono recarsi direttamente in farmacia per il ritiro dei farmaci, possa diventare realtà.

di questo chiarimento che è stato dato, inviterei la senatrice Zampa a ritirare l'emendamento 4.301, proprio per non mettere in imbarazzo l'Assemblea

perché il sostegno che diamo alle aziende che potrebbero essere messe in crisi dal *vulnus* inserito dal *payback* deve essere sanato. Come Gruppo MoVimento 5 Stelle vogliamo essere accanto ai cittadini che soffrono e chiediamo che questo *payback* sia affrontato come misura strutturale.

accetto la riformulazione, anche perché mi fa piacere che il Governo abbia colto l'importanza di questo provvedimento e perché la vostra disposizione ha l'obiettivo di ritardare ulteriormente l'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ambientale e delle foreste in materia di tecniche di preservazione del sughero da organismi nocivi. È stato certificato che la mancata adozione di questo decreto e quindi il mancato trattamento termico del sughero hanno un effetto catastrofico sull'intera filiera del sughero. scelta della maggioranza di ritardare ulteriormente l'approvazione di questo decreto individuo delle motivazioni non economiche e produttive, ma semplicemente politiche. Non capiamo quali siano queste motivazioni diverse da quelle semplicemente economiche e produttive. Il ruolo che dovrebbero avere invece le istituzioni non è tanto ritardare

il *bonus* per lo psicologo a scuola, perché non inerente alla proroga, ma sappiamo tutti quanto bisogno vi

lo *screening* su una platea di persone per individuare eventualmente, la presenza in esse del virus. Ci sono terapie straordinarie che consentono di salvare delle vite umane e, siccome la campagna di *screening* non sta avendo successo, si chiede di prorogare i termini

Il Governo in un precedente provvedimento ha raddoppiato la cifra erogabile per il cosiddetto *bonus* psicologo, riducendo però i fondi a disposizione. Questo vuol dire che riduciamo ulteriormente la platea dei cittadini italiani che possono usufruire di un'assistenza psicologica gratuita o comunque con un contributo dello Stato in un momento di grave difficoltà della popolazione, come tutti abbiamo riconosciuto. Tutti trasversalmente abbiamo presentato emendamenti e parlato a favore delle misure di sostegno psicologico, ma poi riduciamo le somme. Nella passata legislatura, nel corso del 2020, eravamo riusciti a ottenere prima 10 milioni, poi altri 15, per un totale di 25 milioni solo per il 2022

sia per le sedute effettuate in presenza che per quelle da remoto, dal momento che tutti quanti abbiamo visto che ci sono modalità alternative per poter andare incontro ai bisogni di assistenza dei cittadini italiani. Spero davvero che vogliate rivedere la vostra posizione e votare a favore

il rinnovo del personale, chiamiamolo ex Covid, per la scuola. Ecco, c'è l'occasione, così come l'abbiamo fatto noi, di rinnovarlo. Sono certa che Fratelli d'Italia sarà capace di sostenere ciò che in opposizione ci ha chiesto e noi abbiamo sostenuto, e cioè il rinnovo del personale docente e amministrativo, chiamiamolo ex Covid. *(Applausi)*. Le scuole hanno bisogno di personale? (testo 2) e dimostrate che siete per una scuola efficiente ed efficace.

MEF. Vorrei sottolineare che i legislatori dovremmo essere noi e non i tecnici. Ritiro,

i termini, per il Ministero dell'università, per utilizzare le risorse a disposizione della tecnostruttura che abbiamo istituito con la legge di bilancio 2020, che ancora non è partita, perché mancano i decreti attuativi del Ministero dell'università, e che serve alla programmazione del personale medico specialistico. Cosa è successo in questi anni? Noi spesso sentiamo dire che in Italia mancano medici,

ogni anno, solo 6.000 potevano accedere ai corsi di specializzazione. Oggi questo imbuto formativo è stato chiuso, nel senso che si sta colmando, perché i posti per la specializzazione sono 13.400 all'anno. Manca però questo strumento fondamentale, che pure è stato istituito per legge nel 2020. Manca, cioè, l'organismo che ci permette di programmare quali sono gli specialisti che servono. servono. Da un lato, il ministro Bernini ha risposto a una mia interrogazione in Aula dicendo che è volontà del Ministero di far partire quanto prima questa struttura di missione; dall'altro lato, però, non prevede la proroga dei termini previsti per l'utilizzo di queste risorse. E noi temiamo che, se si procede con la lentezza con cui si sta avanzando, vi sia il rischio che i due milioni di euro che sono stanziati ogni anno dal 2020, e che ancora non sono stati utilizzati non essendo la struttura partita, si perdano. Tra l'altro, è stato appena ritirato l'interpello che lo stesso Ministero dell'università ha fatto per la nomina del direttore di questa struttura di missione. Quindi, non capiamo davvero se quella che per noi è una priorità, quella della programmazione del personale sanitario o del personale specialistico medico, lo sia anche per il Governo.

grazie a un lavoro che - lo ripeto - è precario. Se questa è la soluzione che avete pensato per i docenti precari dell'AFAM, mi pare che stiate facendo un errore molto grande, che peraltro

troppa autonomia da parte dei singoli istituti nel reclutamento dei docenti. Voi, in un colpo solo, ignorate la sentenza del Consiglio di Stato e calpestate i diritti dei lavoratori precari dell'AFAM. Peggio di così penso fosse difficile fare. Per questo, vi chiediamo di votare favorevolmente questo emendamento, che vi permette di evitare un grosso errore.

Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno 6.301, che riguarda la proroga di un finanziamento legato alla fondazione Tecnopolo Mediterraneo. un finanziamento di 9 milioni che, qualora non venga prorogato, rischia di far saltare l'iniziativa legata all'istituzione del Tecnopolo Mediterraneo. Chiedo quindi al Governo e alla maggioranza di votare positivamente

il tema dell'emendamento 6.12 sia un'indebita scorciatoia rispetto a quanto dice il Consiglio di Stato; non aiuta a stabilizzare il precariato AFAM, e anzi costringe davvero a

in dichiarazione di voto, unendo il mio intervento a quelli dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto. Signor Presidente, colleghi, qui siamo parlando di uno dei temi più importanti del provvedimento.

uno dei settori che permette al nostro Paese di essere conosciuto nel mondo, che aumenta la nostra credibilità nel mondo; ovunque amano il nostro Paese in virtù della nostra arte, della nostra musica e in virtù di quello che i lavoratori dei nostri istituti musicali e artistici riescono a fare, costruendo nuove generazioni di musicisti e artisti. Sono centinaia e centinaia gli studenti che da tutto il mondo vengono in Italia per studiare nei nostri conservatori e nelle nostre accademie, e qui invece, un emendamento della maggioranza di Governo, surrettiziamente, in un provvedimento che nulla c'entra, colpisce duramente la potenzialità del settore dell'alta formazione artistica e musicale dei conservatori e delle accademie, interrompendo quel percorso importante, virtuoso, che in questi anni abbiamo costruito, di immissione in ruolo di professori nelle accademie, nei conservatori, negli istituti coreutici e musicali. Interrompendo le immissioni in ruolo si dà un colpo a tutta la filiera; non solo vengono mortificate le professionalità di centinaia e centinaia di lavoratori, ma viene anche colpita l'intera filiera. L'emendamento che avete introdotto - e che noi qui chiediamo con forza che venga abrogato - mortifica quei lavoratori, impedisce la stabilizzazione, cancella le graduatorie nazionali, rimanda a non si sa quando. Noi chiediamo invece che siano date subito risposte serie e positive. Chiediamo che continuino le immissioni in ruolo e venga sostenuto questo settore decisivo per la cultura e la crescita del nostro Paese.

ragioni di giustizia sostanziale, anche perché nell'emendamento specifichiamo chiaramente che ci debba essere una valutazione del magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale. Quindi, se a quelle persone è stato è stato garantito un permesso, ne stanno già godendo e stanno rispettando le condizioni che il magistrato di sorveglianza considera valide per continuare a goderlo, non si capisce perché sospenderlo per un approccio di tipo burocratico. L'unica cosa che abbiamo da dire è che è scaduto un termine:

ci sta spiegando, con il suo Ministro della giustizia, che la sanzione penale, la reclusione e la perdita della libertà personale non sono l'unica soluzione. Stiamo sottolineando continuamente, con grande visibilità sui giornali, che la pena deve avere una funzione rieducativa del detenuto. Qui si tratta di detenuti che hanno ottenuto dei benefici, rispetto ai quali stanno rispettando tutte le condizioni. Il Senato della Repubblica, sordo a ragioni di giustizia sostanziale, dice che

che risponde a ragioni di giustizia sostanziale e non crea alcun allarme sociale, perché quelle persone sono già nel regime di semilibertà, e quindi non hanno creato una condizione di pericolo rispetto all'ordine pubblico e alla tranquillità sociale, qual qual è la ragione sostanziale di una tale scelta. Mi rifaccio ai valori della nostra Costituzione, che ci accomunano tutti. Con quale faccia e con quale spirito diciamo loro di rientrare in carcere solo perché è scaduto un termine?

Abbiamo già discusso di questo tema in Commissione e in Assemblea e mi scuso con i colleghi se torno a riproporlo, ma

che sono state sperimentate durante la pandemia. Durante la pandemia, anche per affrontare il drammatico tema del sovraffollamento delle carceri, il Governo, con un decreto-legge, ha introdotto due misure alternative alla detenzione in carcere, che - come ricorderete prorogate anche in occasione del precedente decreto milleproroghe. Queste due misure alternative si rivolgono rispettivamente a coloro che già godono di licenze o permessi premio straordinari e ai detenuti in regime di semilibertà di semilibertà o che devono scontare pene residue inferiori ai diciotto mesi, esclusi naturalmente i reati di maggiore gravità sociale. Nei confronti di queste fattispecie, il Governo, durante la pandemia, ha introdotto due misure

alla fine del 2021, il Parlamento decise di prorogare ulteriormente di un anno, fino al 31 dicembre 2022, queste due misure. I dati che ci ha fornito il Ministero confermano che si tratta di misure ragionevoli, che non hanno destato alcun allarme sociale e non hanno visto, neanche nel 2022, un solo caso

a voi, colleghi, cos'è il PNRR e cosa è successo, anche a livello comunitario, in conseguenza di ciò che la pandemia ci ha fatto sperimentare.

sentire da parte del Governo l'indisponibilità a considerare questa proposta.

Il tema non è il fatto che è scaduto un termine, ma che non c'è più la pandemia. Queste misure si fondavano esclusivamente su una ragione che è venuta meno; poi, quando sarà quando sarà il momento e quando si affronterà questo tema in modo organico, si potrà ragionare sulle misure alternative, ma queste misure alternative sono fondate sulla pandemia che, per fortuna, è venuta meno. Soltanto questa è la ragione per la quale in questa sede il parere dei relatori (e presumo anche del Governo) è contrario.

il rischio che si corre non prorogando questa misura. La questione non riguarda la presenza o meno della pandemia; la questione è che ci sono detenuti che in questo modo vengono riportati indietro, nonostante abbiano dato buona la prova di sé nel trattamento e nel percorso riabilitativo. Questo è il principio che sta dietro a questa norma.

perché vorrei chiedere subito l'intervento in Aula del ministro Schillaci, affinché ci comunichi una notizia straordinaria di cui non mi ero accorta, cioè che è finita la pandemia. *(Applausi)*. È una notizia a cui tutto il Paese guardava con grande

del detenuto non può essere mutato e interrotto nella sua continuità. Pertanto, chiediamo vivamente al Governo e ai relatori di rivedere fortemente la loro opinione ed il loro parere su questo emendamento.

Voglio ricordare che riportare in carcere persone che hanno ristabilito contatti con la famiglia e con la società e che si sono avviati verso un percorso di redenzione è una violenza gratuita.

Balboni. Il 31 dicembre 2022 non si è verificato qualcosa di significativo relativamente alla pandemia. Come stavamo il 31 dicembre 2022, stiamo il 1° gennaio 2023. Non si capisce allora per quale motivo i detenuti che hanno ottenuto dei permessi premio e che hanno avuto delle condizioni trattamentali che

concittadini che hanno usufruito della possibilità di rientrare in un circuito virtuoso dentro la società e abbiamo detto loro, con una ragione puramente burocratica,

come il Governo e come il Parlamento possano dirlo a queste persone. Tra l'altro, siamo tutti d'accordo che le carceri sono un luogo criminogeno. Molti dicono che il carcere sia l'università del crimine. Che interesse abbiamo, come società, di riprendere persone che non hanno compiuto alcun reato in quel periodo? Persone il cui destino comunque colleghiamo alla valutazione del magistrato di sorveglianza. Non c'è alcun automatismo, ma ogni caso viene verificato. Invece noi che cosa facciamo? Indipendentemente

che abbiamo messo in opera, al fatto che abbiamo violato, a mio avviso, un principio costituzionale e impegna il Governo quantomeno a trovare delle soluzioni razionali per evitare che il mero passaggio del tempo produca effetti giuridici, sociologici e umanitari che sono francamente incomprensibili. Chiedo quindi ai colleghi di votare a favore del mio ordine del giorno.

Credo però che le parole del relatore siano sincere e devo dire che anche in Commissione il Governo è venuto a dire di non essere riuscito, né con il precedente provvedimento legato alla legge di bilancio, né adesso con il milleproroghe, ad approvare un emendamento come quello presentato dal senatore Scalfarotto o quello presentato dal senatore Giorgis e da altri,

Presidente del Parlamento europeo dal 1997 al 1999, è stato a lungo vice presidente e presidente della commissione affari costituzionali, ma soprattutto è stato un grande democratico cristiano e un grande amico dell'Italia. Ha servito il suo Paese, la Spagna, come ambasciatore in Italia; anche nel corso del suo mandato di Presidente del Parlamento europeo non sono state poche le occasioni in cui ha mostrato interesse, ammirazione e stima

Visto che c'è una richiesta di sospensione di venti minuti o mezz'ora e visto che nel pomeriggio abbiamo fissato il Consiglio di Presidenza, per poter dare corso all'ampliamento del numero dei senatori Segretari, così come richiesto

La ringrazio, Presidente. A nome del Gruppo Forza Italia, saluto con grandissima soddisfazione la sentenza di assoluzione del presidente Berlusconi, perché il fatto non sussiste. anni di processo, più di 600 udienze, milioni di euro spesi a carico dei contribuenti, una gogna mediatica, giudiziaria e politica che richiedono una profonda e strutturale riforma della giustizia per la tutela di tutti i cittadini, anche quelli che non hanno le possibilità e gli strumenti per difendersi. Questa sentenza ristabilisce la verità, ma non restituisce il danno di immagine provocato

né permette al presidente Berlusconi di sanare la grave lesione dell'onorabilità e della reputazione della sua persona e della forza politica che rappresenta.

La domanda è chiara: sentite di assumervi la responsabilità di non permettere a queste persone di avere un piatto di pasta ogni giorno per sé

ieri, che i lavoratori, quando si è alla fine di un processo, sono quelli che pagano di più, soprattutto quelli con ridotte capacità produttive. Che il Parlamento non trovi un milione di euro per coprire la cassa integrazione dei lavoratori di Termini Imerese credo che sia una vergogna e per questa ragione chiedo di approvare

10.302. Si tratta di una norma che estende un finanziamento che è stato previsto soltanto per

due anni che l'intera Regione è bloccata, lo sappiamo noi liguri, ma lo sanno tutti coloro che devono passare attraverso le nostre autostrade. Di fronte a questo, sarebbe necessario un intervento urgente per ripristinare la possibilità per tutti i cittadini di utilizzare le autostrade. C'è bisogno di una forte spinta del Governo perché la società decida a cantierare in maniera compatibile con la vita di tutti i cittadini e con la sicurezza che le infrastrutture, soprattutto nella nostra Regione, richiedono. Di fronte a questo, invece, è scattato l'aumento automatico dei pedaggi. Noi riteniamo che sia fondamentale dare un segnale ad Autostrade, almeno bloccando l'aumento dei pedaggi per far sì che arrivi il messaggio chiaro che devono essere ripristinate al più presto le vie di comunicazione. Per questo chiediamo di prorogare il termine richiesta da genovesi che non vogliono pagare il pedaggio, ma è l'unico modo che abbiamo per fare pressione rispetto a una situazione che è obiettivamente insostenibile. Chiediamo che la società Autostrade non possa applicare l'aumento dei pedaggi. Credo che non sia una questione

Per lo stesso senso istituzionale, le chiedo di non polemizzare; è rispetto per l'Assemblea e senso delle istituzioni

La seduta è aperta

siamo arrivati

molta parte quantomeno dell'opposizione è contraria a qualsiasi tipo di attenzione nei confronti delle esigenze dei balneari, perché magari vogliono le gare immediatamente, senza dare il tempo a

non dovrebbe negare la necessità di un tavolo tecnico consultivo, proprio per stabilire i passaggi, qualunque essi siano:

ma a maggior ragione se si ritiene si debba andare verso una radicale trasformazione delle dinamiche di questo settore, che sarebbe determinato da un'immediata applicazione della cosiddetta norma Bolkestein. Ecco perché il nostro

pregiudizialmente contrari a qualunque esigenza di questa categoria, allora si deve votare a favore di questo emendamento, altrimenti pensiamo sia corretto votare contro.

Lei giustamente ha accolto la proposta di sospensione dei lavori di quest'Aula sulla base di un'istanza che proveniva dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale ci aveva ci aveva preannunciato modifiche ad emendamenti già approvati o addirittura l'aggiunta di emendamenti nuovi rispetto al lavoro delle Commissioni referenti. Non possiamo, per rispetto del Parlamento e per la funzione che ricopre, riprendere questa seduta senza chiarirci sulle ragioni di questa sospensione. Il Ministro ci deve spiegare non solo cos'è successo, ma siccome parliamo di un tema molto delicato, perché qui stiamo parlando di concessioni balneari, di sentenze già in atto e del rischio di sanzioni e di potenziali ricadute anche sulla finanza pubblica: noi abbiamo bisogno della trasparenza. È stata scelta da parte della maggioranza una strada a nostro avviso fin qui sbagliata, non coerente con i princìpi fondamentali e le regole della finanza pubblica: noi abbiamo bisogno di capire cos'è successo e quali erano le ragioni alla base di questa sospensione. Ministro Ciriani, se lei ritiene può intervenire, perché in effetti lei ha chiesto una sospensione.

Signor Presidente, accolgo la richiesta del collega Manca per dire che avevo chiesto una sospensione per verificare se c'era la necessità di un approfondimento su alcuni emendamenti già depositati e non ancora votati, la possibilità di aggiungere altri emendamenti, perché sono giunte richieste da alcuni Ministeri per ulteriori testi normativi e anche per la verifica ulteriore su alcuni emendamenti. Abbiamo fatto le verifiche del caso e non c'è necessità di modificare alcunché sul testo depositato, né aggiungeremo altri testi

abbiamo avuto la sensazione netta che la motivazione

Signor Presidente, con assoluta trasparenza, il tema dei balneari è un tema su cui il Governo ci ha chiesto un approfondimento, ma non c'è nulla da nascondere. un approfondimento e una valutazione attenta, su una questione politica di cui si discute da tempo e di cui si è discusso anche nel precedente Governo. Quindi, con estrema chiarezza, c'è stato un confronto in maggioranza e quest'ultima ha deciso di andare avanti e vi spiego anche perché.

una volta per tutte. La direttiva Bolkestein dice che bisogna andare a gara se la risorsa è considerata scarsa: questa è la direttiva. Chiedo a

che in vent'anni ha tentato di mettere in campo questa mappatura, per capire effettivamente se la risorsa è scarsa o no, è stato il senatore e allora ministro Gian Marco Centinaio, con la legge n. 145 del 2018!

interessi, le applichiamo sempre nel modo più restrittivo possibile, perché noi siamo per l'Europa ed è l'Europa che ce lo chiede, è l'Europa che ce lo dice, è Bruxelles che ci chiede di intervenire ed è arrivato il commissario... *(Applausi)*. Questo atteggiamento servile

Con la sentenza del Consiglio di Stato, intanto, però, se facciamo la mappatura e verifichiamo se la risorsa è davvero scarsa, si può aprire un'interlocuzione con l'Europa per vedere se effettivamente la direttiva Bolkestein interviene sul nostro territorio così come si è detto in tutti questi anni. Questo è stato il ragionamento che avevamo chiesto al Governo Draghi; non siamo riusciti a ottenerlo, abbiamo dovuto mediare perché eravamo in un Esecutivo di unità nazionale, quindi siamo arrivati alla soluzione

se abbiamo un po' di tempo per fare una mappatura, poi se risulta che la risorsa è scarsa bisognerà fare le gare; c'è già una legge, vareremo i decreti attuativi e si farà quanto necessario. Perché negarci a priori la possibilità, una volta per tutte nel 2023, con gli strumenti che abbiamo,

penso però che questa possa essere una soluzione, anzi un ottimo trampolino di lancio per il Governo per andare in Europa a fare queste verifiche. In conclusione

che la questione sollevata dalla collega Paita sia emersa con un elemento di verità, cioè che in sostanza c'è stato un tema, si è passati dal parlare sull'ordine dei lavori su un tema di tipo procedurale. PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, quindi?

Se ha il microfono spento io non la sento, lo capisce? Chiede di parlare di nuovo sull'ordine dei lavori? dei lavori? Si accomodi, è agitato. Intervenga sull'ordine dei lavori, purché non sia lo stesso identico ordine dei lavori che abbiamo appena affrontato.

ha sostenuto l'estensione delle concessioni al 2024. A quelli che si scandalizzano dico che già la legge del Governo Draghi prevedeva, qualora i Comuni avessero riscontrato problemi, che la la procedura si potesse estendere al 2024 e non concludersi entro il 2023. Dopodiché abbiamo chiesto comunque un'estensione delle concessioni perché non ci risulta né concluso il monitoraggio né chiarita la situazione. Il Gruppo Lega con un emendamento del senatore Marti e del capogruppo Romeo, che ho avuto anch'io l'onore di firmare, invita a fare il monitoraggio in un determinato tempo o a costituire un tavolo che possa verificare con tutti i Ministeri e l'organizzazione che cosa si debba fare. Vi sono poi altri emendamenti anche dei relatori che, in un concorso di tutte le forze politiche del centrodestra, hanno chiesto di estendere il tempo per il monitoraggio ed evitare che i Comuni facessero delle gare in questa fase.

decisioni del Consiglio di Stato, ulteriori decisioni annunciate dalla Corte di giustizia europea, ma anche ricorsi del TAR di Lecce che difende i balneari, la direttiva Bolkestein che per noi riguarda

però gestite dai Comuni; non le spiagge abbandonate che diventano una discarica. Non vogliamo le spiagge libere dove non c'è il bagnino, si affoga se non c'è il soccorso e si trovino solo detriti portati dalle mareggiate. La spiaggia libera è una spiaggia gestita da un Comune, non è una spiaggia abbandonata. Noi tuteliamo le imprese italiane e diciamo all'Europa che deve cambiare indirizzo; l'abbiamo fatto tutti nel centrodestra. Poi si sono tentate, Presidente, mediazioni e valutazioni, la cosa è complessa. Mi pare che ci sia la volontà di dire alle autorità europee che devono valutare diversamente la questione. Io me ne occupo da molti anni. Non vedo oggi il senatore Monti, ma lo dico pubblicamente e non mi potrà smentire: quando lui era Presidente del Consiglio e io ero Capogruppo, gli andai a spiegare, con una cartina dell'Europa, che in Italia le spiagge sono una risorsa del turismo, mentre in altre parti d'Europa ragioni climatiche non le rendono tali. C'è una specificità italiana, che noi difendiamo; vogliamo tutelare le imprese, che sono spesso piccole imprese familiari. E a quelli che, alla Giavazzi, hanno ispirato male anche l'azione di altri Governi diciamo di andare a vedere adesso, a febbraio, quelle aziende balneari distrutte dalle mareggiate, dalla Liguria alla Calabria, dal Veneto alla Puglia. Chi risarcisce queste imprese fragili, esposte all'erosione delle coste, alle mareggiate, a danni di mille maniere? *(Applausi)*. Ma di cosa parliamo? Allora parlate con questi lavoratori del mare e della spiaggia, Ministro, perché il mare poi comincia dopo la spiaggia. Noi li difendiamo con convinzione, consapevoli, Presidente, che c'è un contenzioso,

Si paghi il giusto, si rispetti l'ambiente, ma si rispettino anche le imprese. Sono convinto che il Governo, in tutte le sue componenti (sono vari i Ministri che se ne devono occupare, dal mare alle infrastrutture, al turismo, agli affari europei, all'ambiente), difenderà le imprese italiane. Noi lo facciamo nell'Aula del Parlamento e, se il Consiglio di Stato sbaglia, noi non vogliamo sbagliare come il Consiglio di Stato.

abbiamo sentito due cose leggermente diverse nei due interventi di maggioranza. Da un lato il senatore Romeo, giustamente, dice che serve il monitoraggio per capire se la risorsa è scarsa; dall'altra parte il senatore Gasparri, che ha già la verità, dice che la risorsa non è scarsa e che quindi forse non serve fare monitoraggio. Fuori di battuta, per il suo tramite, Presidente, mi rivolgo al presidente Romeo per ringraziarlo del suo intervento. Essendo una persona perbene e seria, che non ha mai fatto interventi ipocriti in quest'Aula, egli ha detto esattamente le cose come sono andate. descritto quello che è successo in quell'ora di sospensione e credo sia giusto ringraziarlo per l'onestà intellettuale con cui è intervenuto. Egli ci ha fatto capire, però, che alcuni problemi c'erano e che non è dato sapere, da parte delle opposizioni, come sono stati risolti e perché improvvisamente sono spariti. Alcuni elementi problematici provo a dirli io. Certamente il tema dei balneari, in particolare per il nostro Paese, che ha 8.000 chilometri di costa, è un tema complicato e complesso, che non ha una soluzione facile. Vent'anni di dibattito su come risolvere questo problema hanno portato a una soluzione che ancora non c'è, perché il problema è complesso e perché ci sono tantissimi imprenditori seri che hanno investito e che hanno il diritto di continuare le loro attività. Ci sono però anche alcuni, pochi, imprenditori un po' meno seri, che potrebbero vedere con favore una proroga *sine qua non* dei provvedimenti di concessione rispetto al tema della Bolkestein, perché continueranno a fare quello che non hanno fatto, cioè a non investire e a sfruttare le nostre coste pagando praticamente zero. Credo che questo sia il tema più rilevante da affrontare. Credo, invece, che l'equilibrio che avevamo raggiunto in un Governo di unità nazionale nella scorsa legislatura, che aveva portato ad un testo molto discusso, che aveva visto tutte le forze politiche contribuire, retrocedendo da alcune posizioni per individuare tutti assieme la soluzione più condivisa possibile, fosse da mantenere. Ed è per questo che c'è il mio emendamento abrogativo. Io non abrogo qualcosa che avevamo previsto nella scorsa legislatura, al quale la mia forza politica aveva partecipato attivamente; semplicemente, abrogo delle modifiche che ritengo non sia il momento di fare. Sul dibattito in Commissione, è evidente che le forze di maggioranza hanno proposto e poi approvato dei testi emendativi. Noi avremmo preferito, come forze di opposizione (e lo abbiamo detto in tanti momenti) che ci fosse un unico testo del Governo, sul quale vedere espresso un parere certificato da una bollinatura e da una relazione tecnica, che non c'è, rispetto ai profili finanziari di quello che stiamo facendo. È evidente, infatti, che prorogare il tema delle concessioni porta a un minor gettito potenziale. Se infatti avessimo fatto il lavoro in questa annualità, avremmo potuto iniziare un incremento degli oneri concessori, che avrebbero portato a più risorse dello Stato. Giusto o sbagliato

(a nostro avviso, più che eventuale, certa) procedura di infrazione, che certamente avrà un impatto finanziario sulle casse dello Stato. Anche da questo punto di vista, noi non abbiamo nessuna certezza. Io mi chiedo, quindi, con quale forza questo provvedimento esca da quest'Aula avendo la garanzia che non ha una incidenza sui profili finanziari del bilancio dello Stato. Per questo motivo noi presentiamo un emendamento abrogativo di una parte delle proposte della maggioranza. Torneremo sull'argomento con l'ultimo emendamento, di cui discuteremo prima dell'emendamento di coordinamento, perché anche su quel fronte ci saranno alcune considerazioni da fare. Io ritengo di poter insistere per un intervento chiarificatore da parte del Governo in questo momento rispetto alla procedura di infrazione e rispetto agli oneri finanziari, che l'approvazione degli emendamenti già approvati in Commissione anche in quest'Aula potrà produrre sulle casse dello Stato.

vorremmo invitare anche i colleghi della maggioranza ad una riflessione approfondita su quanto stiamo discutendo. Noi abbiamo avuto, lo voglio ricordare, una sospensione di un'ora dei lavori di questa Assemblea, chiesta dal Governo. Che ci siano problemi è stato ammesso da un autorevolissimo esponente della maggioranza, nella figura del senatore Romeo; problemi che però non sono stati dettagliati, come secondo noi andrebbe fatto, da parte del Governo.

una sentenza del Consiglio di Stato di una durezza e di una nettezza senza precedenti; incrocia delicate problematiche di normativa europea e incrocia anche l'attuazione del PNRR, all'interno del quale il tema della concorrenza è una delle riforme più significative. Io vorrei ricordare al Governo e ai colleghi della maggioranza che vi è già stata una retromarcia da parte del Governo sul tema del POS, che, mi sia consentito dire, ha una valenza

al di là dell'orientamento di ognuno di noi sulla vicenda dei balneari, perché abbiamo il diritto di sapere se ci sono dei profili di criticità dal punto di vista della copertura, degli oneri, del contenzioso e dell'attuazione o meno del PNRR, in relazione al mantenimento o meno della proroga di un anno che è stata approvata in Commissione Noi dobbiamo decidere con la pienezza delle informazioni, cui abbiamo diritto nel momento in cui andiamo a votare su una tematica di enorme importanza, che riguarda decine di migliaia di operatori, interessi economici molto rilevanti e, nella sua delicatezza, il rapporto di questo Paese con la Commissione europea per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

che hanno investito e per le quali il lavoro come balneare rappresenta l'introito prevalente, se non l'unico.

ma qui non stiamo parlando di questo. Qui stiamo vendendo una finta proroga; stiamo dicendo agli operatori che forse c'è del tempo in più per arrivare alle gare, e mentre non facciamo gli interessi di una parte, facciamo il danno dell'Italia mettendo a repentaglio le risorse del PNRR. *(Applausi)*. Vorrei poter sostenere lo abbiamo fatto in passato - che servono le definizioni e che in qualche modo c'è un aspetto tecnico che ci fa richiedere tempo. La Commissione europea ha già respinto perché, come ha detto il collega Patuanelli prima, non è una risorsa scarsa. Quindi, quella non è una motivazione plausibile. E allora come si fa quando si prova a difendere l'interesse generale? Da un lato, non si possono raccontare balle ai balneari *(Applausi)*, e dall'altro lato, non si può responsabilmente mettere a repentaglio le risorse del PNRR. Abbiamo a che fare con un Governo che vende modifiche al PNRR che non si capisce quali siano e al tempo stesso si sa che, come è accaduto sulla delega fiscale, come avvenuto sulla concorrenza e come rischia di accadere sui balneari, questi tre punti sono per la Commissione europea europea fondamentali per confermare le risorse del PNRR, senza le quali questo Paese ha un danno molto più ampio di una finta proroga. Ecco perché invito la maggioranza a fare quantomeno gli interessi del Governo: se volete aiutare Giorgia Meloni, se volete sostenerla in Europa, fate in modo che l'emendamento non passi. Dite la verità ai balneari: li abbiamo aiutati finché si è potuto, ma è venuto anche il momento di dire sì alle gare e soprattutto di dire sì ai fondi del PNRR, senza mettere a repentaglio risorse

è giusto che una maggioranza politica si assuma la responsabilità, ma allora smettetela di fare sceneggiate. Dite che politicamente avete deciso di fare una cosa, assumetevene la responsabilità, e basta.

in relazione alla confusione che si è verificata in Aula quest'oggi, se nel frattempo ci sono state delle interlocuzioni tra il Governo

giorno fosse accolto, perché il Governo ha il dovere di coinvolgere all'interno di questa discussione tutti gli operatori. È corretto, sono operatori che hanno i loro interessi, ma in realtà il demanio fa parte di un intero comparto turistico, che fa riferimento agli albergatori, agli operatori e ai lavoratori di tutta l'area turistica. Soprattutto,

sul tavolo che viene portato avanti in questo momento, che esclude completamente dalla discussione tutti i cittadini, tutti coloro che operano nell'ambito delle spiagge, tutti coloro che lavorano in quel comparto e tutti quelli che hanno competenza in materia. Noi abbiamo portato avanti un grandissimo lavoro

contro l'ordine del giorno G10-*quater*.300, per un semplice motivo: il MoVimento 5 Stelle, Presidente, da un lato presenta un emendamento per sopprimere il tavolo, dall'altro lato presenta un ordine del giorno per aggiungere gente al tavolo. Facciano pace con se stessi. *(Applausi)*. Se la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, alla fine noi votiamo contro tutto.

Signor Presidente, vorrei ancora una volta rivolgere un appello al Governo e anche ai colleghi della maggioranza per rivedere il parere contrario su questo emendamento. Stiamo discutendo di dismettere delle società società partecipate che fanno utile. Chiediamo semplicemente una proroga di un altro anno, perché parliamo di aziende sane,

Thiene è uno dei gioielli nazionali che potrebbe finire per essere svenduto a privati, insieme ad altre decine e decine di società partecipate pubbliche, che - insisto - fanno utile e fatturato. Quindi, chiediamo con gran forza di rivedere il parere contrario da parte del Governo, anche perché non si capisce la *ratio* della bocciatura di questo emendamento, non c'è

per i soggetti impegnati nell'area del dilettantismo».

in tanti in maniera trasversale. Si tratta di dare la possibilità alle persone con disabilità di praticare l'attività sportiva grazie all'erogazione di protesi, ausili e dispositivi di tecnologia avanzata oggi non previsti dallo Stato. Sostanzialmente l'ordine del giorno, per il quale mi sarei aspettata un parere favorevole a a prescindere, senza raccomandazioni, chiede di rifinanziare un fondo che ha visto finalmente la sua luce lo scorso dicembre, dopo tre anni di dibattiti, proprio perché è sperimentale e consente di guardare a quelle voci non come spesa, ma finalmente come investimenti. *(Applausi)*. Nel momento in cui noi ci vantiamo di votare trasversalmente l'inserimento dello sport in Costituzione

preferito un parere nettamente favorevole. Tenevo a condividere questa osservazione anche con i colleghi dell'Aula perché siamo tutti coscienti e consapevoli del motivo di questo ordine del giorno. Accolgo poi la riformulazione dell'ordine del giorno

nei limiti delle risorse disponibili, si possa accogliere l'ordine del giorno e il Governo e i relatori possano rivedere la loro posizione. Non mi sembra un argomento che possa mettere in crisi le nostre finanze. *(Applausi)*.

Si tratta del risanamento della città di Messina dalle baraccopoli e della sostituzione della figura del commissario, essendo stato nominato il Presidente della Regione Siciliana; si prevede inoltre la nomina di un subcommissario. Insisto a chiedere che sia il sindaco di Messina a essere nominato subcommissario o, in alternativa, che l'incarico di subcommissario, visto che sembra che il Governo ci tenga tanto a darlo a un soggetto privato e non a una carica istituzionale, sia a titolo gratuito. Non capisco perché

sull'emendamento 18.304, perché il risanamento non è semplicemente comprare alloggi dove trasferire le persone che vivono nelle baracche del Comune di Messina, ma è anche un'opera di riqualificazione ambientale e urbanistica, per la quale ci sono progetti importanti già finanziati dal Comune di Messina. Spogliare il Comune dei fondi, per farli entrare in una gestione in capo solo al commissario, al quale si dice che deve privilegiare l'acquisto di alloggi, è una misura iniqua ed è soprattutto una misura contro lo stesso territorio di Messina.

che conoscono benissimo la Sicilia e conoscono Messina. Si tratta di una città che è stata bistrattata e dimenticata. Noi invece ce ne siamo occupate, e parlo anche alla sottosegretaria Siracusano. Adesso, sinceramente, togliere il commissariamento al prefetto o non darlo al sindaco e darlo invece in mano al vostro Presidente di Regione, con l'ansia di un asso pigliatutto, riteniamo che sia un'offesa alla città.

questa vicenda, di cui si era già occupato il precedente Governo e che riguarda Messina, effettivamente non si comprende per quale ragione debba esserci una inversione di *governance* in questo momento, peraltro con oneri aggiuntivi a carico dello Stato e all'interno di un provvedimento rispetto al quale la battaglia sugli oneri è stata particolarmente importante, anche in Commissione bilancio. Quindi, aderiamo con forza a questo emendamento e ci auguriamo che anche i colleghi siciliani della maggioranza si uniscano a questo tipo di proposta.

Signor Presidente, torniamo sul tema di cui abbiamo ampiamente dibattuto questo pomeriggio, riguardante gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione e a questo punto anche in Aula, ossia le concessioni demaniali. Come è noto, la legge n. attraverso tre articoli di legge, tratta di tre fattispecie interconnesse ma diverse: da un lato, la questione del monitoraggio del disegno delle attuali concessioni in essere, della plastica evidenza di ciò che accade sui territori delle coste italiane; dall'altra parte, il dispositivo determina le normative rispetto alle concessioni in essere, cioè fino a quando potranno essere prorogate e fino a quando i Comuni potranno intervenire con i bandi. All'articolo 4 vi è poi il cuore della legge delega in materia di concessioni balneari, poiché il comma 1 di quell'articolo interviene delegando il Governo, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo e in coerenza con la normativa europea, ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 118 del 5 agosto 2022

sottostare ai dettami del comma 2 dell'articolo 4, cioè tutto quell'impianto complessivo di principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione. Governo e maggioranza sono intervenuti su questi testi, come noto, attraverso tre fattispecie emendative: il Gruppo Lega ha istituito il tavolo, stabilendo un primo regime di proroga; poi, sono intervenuti l'emendamento Ronzulli di Forza Italia e quindi l'emendamento del Governo, che hanno spostato data e termini di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e parzialmente all'articolo 4. Nessuno è intervenuto sulla proroga relativa alla legge delega rispetto al cuore della normativa. Mi verrebbe da dire che qui casca l'asino, nella misura in cui si manifesta

perché dovrà essere fatta una nuova legge delega nei confronti del Governo che avrà nuovi criteri e nuovi tempi di attuazione. Quindi, non si arriverà al 2024, ma al 2028;

la mia forza politica e mi sembra di capire le opposizioni riteniamo che questo ci esponga a un rischio di infrazione enorme. Per risolvere questo tema abbiamo presentato un emendamento che sposta i termini della legge delega: da termine entro ottobre di quest'anno, in modo da poter esercitare quell'esercizio di delega, dopo aver fatto il monitoraggio, dopo aver istituito il tavolo, dopo aver determinato se le spiagge sono o no un bene ancora disponibile o se sono troppo poche, come qualcuno dice, o sono troppe, come dice qualcun altro. In questo modo risolvete anche il tema della legge delega, e qui si vedrà la reale volontà di Governo e di maggioranza.

visto che nella legge sulla concorrenza, all'articolo 2, è previsto il tema della mappatura, in attesa di capire, tramite la mappatura, se la risorsa sia scarsa o meno, si prende un po' più di tempo sulla delega e nel frattempo si prorogano i termini per dare anche la possibilità di intraprendere questa interlocuzione con l'Europa, che è giusto che un nuovo Governo politico intraprenda.

messo a punto il discorso sulle concessioni balneari a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato. Allora c'era il ministro Garavaglia Garavaglia e, per evitare che venissero sequestrate le spiagge dei nostri balneari, si fece quel tipo di intervento. Poi le mediazioni fanno parte ampiamente del discorso della politica. Però chiariamo una volta per tutte

del PNRR dall'Europa: lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Nuyts, smentendo così una *fake news* ripetuta troppo spesso dalla politica e dai *media* generalisti. Mi scusi, senatore Misiani, ce lo dice l'Europa. Presidente, quando parliamo di Europa, penso che tutti noi conosciamo la differenza tra la Commissione europea e la Corte di giustizia europea, e qual è la gerarchia in termini di autorità. C'è una sentenza, la Promoimpresa, che è chiarissima

che non è chiaro negli interventi che ci sono stati), sono soggette a forme di selezione e - questo non c'entra con la specifica vicenda dei balneari, ma fa parte di tutte le risorse scarse, ad esempio quelle dello spettro radio, come sappiamo - devono essere soggette a procedure selettive. Tali procedure certamente sono in funzione della scarsità, che non è soltanto fisica ma anche di mercato. Su questo ci siamo, ma il punto è che assegnazioni che non prevedano queste valutazioni sono comunque esse stesse illegittime. L'argomento che è stato qui ribadito e che ho sentito, ossia che in assenza di valutazioni della scarsità le attuali assegnazioni sono legittime, va capovolto: in assenza di quella valutazione, qualunque assegnazione che non abbia un criterio selettivo è illegittima per definizione. *(Applausi)*. Quindi facciamo attenzione dal punto di vista della costruzione giuridica. Quando parliamo di concorrenza e di tutela del consumatore, guardiamo anche agli interessi delle attuali piccole imprese: ma perché non devono essere nella vostra mente? Parliamo delle vincitrici di gare e di selezioni competitive: perché non dovrebbero essere loro le prime aggiudicatarie di questi processi trasparenti che l'Europa ci chiede non solo nella tutela

togliere la questione dei balneari dalla propaganda elettorale e riportarla in un alveo che è quello delle decisioni che hanno assunto anche le massime istituzioni del nostro Paese. In quest'Aula ho sentito diversi esponenti della maggioranza dire che va riformata la sentenza del Consiglio di Stato e qualcuno dire che invece va applicata. Quindi anche in questo c'è un tema di interpretazione su cui la maggioranza forse dovrebbe chiarirsi le idee. In ogni caso, su questo tema la discussione che è stata fatta va al di là del caso specifico. Quale Quale rapporto vogliamo avere con le normative e con le istituzioni europee? O crediamo che siano anche le nostre istituzioni, anche le nostre normative, e informiamo tutto tutto il nostro impegno legislativo in una coerente azione, oppure prendiamo una strada che oggi riguarda i balneari, domani riguarderà qualche altra cosa, ma che ci porta lontano non solo dall'Europa, ma dalla credibilità del nostro Paese.

indennizzo risparmiatori) l'Europa non abbia niente da dirci e lo spiego sotto un profilo strettamente tecnico: le somme che compongono il fondo del FIR provengono dai conti dormienti delle banche. Dopo la sentenza Tercas della Corte di giustizia europea, quella che è intervenuta sui presunti aiuti di Stato alle banche, è ben chiaro che i fondi che provengono dal mondo bancario - e questi sono fondi che provengono dal mondo bancario e sono stati finalizzati proprio al ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche - non sono aiuti di Stato. Quindi, su questo tema non ci deve essere interlocuzione con l'Europa, perché è fuori posto. posto. Da questo punto di vista, ringrazio il Governo che ha recepito questa mia osservazione di natura tecnica. Abbiamo la possibilità di dare una risposta ulteriore ai risparmiatori truffati dalle banche e su questo c'è stato un impegno *bipartisan* di tutti i nostri segretari di partito durante la campagna elettorale, tant'è che ho molto apprezzato il fatto che il mio ordine del giorno nel frattempo

che sono stati truffati dalle banche abbiano quest'ulteriore ristoro che gli spetta alla luce della legge di bilancio del 2019 e dei principi ad essa ispirati. *(Applausi)*.

quella del collega Paganella e della collega Erika Stefani. Molti conoscono la storia dei truffati dalle banche. Sono persone semplici,

il fondo prevedeva solo 100.000 euro, ma siamo riusciti a portarlo a 1,5 miliardi di euro e siamo riusciti a dare una risposta a 140.000 risparmiatori. Con l'ordine del giorno in esame chiediamo al Governo di procedere all'incremento della percentuale di indennizzo, perché è semplicemente un atto di equità e di aiuto a queste persone che sono state truffate che, giustamente, devono essere ricordate e aiutate dal Parlamento. Quindi, aggiungendo la firma, esprimo anche il nostro parere favorevole. Signor Presidente, anche io intervengo brevemente per sottoscrivere

che prevedeva appunto l'aumento delle risorse del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) e anche l'aumento dei tempi tecnici per verificare ulteriori misure volte a garantire tutti gli aventi diritto ad un rimborso. Qui si sta parlando di indennizzi a favore di risparmiatori e di azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte delle banche, banche, che sono state poste, come ricordato, in liquidazione coatta. Quindi si tratta di un intervento che va nella direzione giusta e che abbiamo più volte sollecitato nel corso di questi anni. Mi auguro che dal voto dell'Assemblea possa essere determinato anche un impegno serio del Governo, affinché questo problema possa essere risolto e affinché tutti i risparmiatori che hanno subito un danno abbiano il giusto rimborso.

che condivide questa battaglia. Crediamo sia giusto risarcire persone che sono state ingannate nella sottoscrizione di titoli, dei quali non conoscevano correttamente il contenuto. Aggiungo che probabilmente c'è stato anche qualche errore, di qualche Governo passato, che forse ha sottovalutato la situazione anche per compiacere l'Europa. Il Gruppo Fratelli d'Italia chiede pertanto di aggiungere la firma dei suoi componenti. Ringrazio il collega e anche il Governo, che nella riformulazione ha tenuto conto delle osservazioni importanti che sono state fatte:

una discriminazione che è in corso, in quanto nell'ambito dell'utilizzo di questo Fondo, con cui andiamo a risarcire i risparmiatori di alcune banche, prettamente le banche venete e del gruppo veneto,

un emendamento per estendere anche a questi risparmiatori la possibilità di accedere al risarcimento. Anche loro sono stati infatti truffati, nell'ambito delle truffe bancarie.

avvenendo e visto che siamo tutti d'accordo, forse il Governo dovrebbe fare uno sforzo in più e anche indicare tempi molto ristretti per fare questa istruttoria tecnica e arrivare finalmente a una soluzione.

per sua natura, è difficile da riassumere e illustrare in pochi minuti. È un testo che interviene in diversi ambiti della vita di cittadini, famiglie e imprese. Il Paese oggi si sta faticosamente lasciando alle spalle l'emergenza sanitaria del Covid. Prima della pandemia, secondo il Censis, 19,6 milioni di italiani

Prima della pandemia, secondo il Censis, 19,6 milioni di italiani sono stati costretti a rinunciare a una visita medica o ad un controllo a causa, purtroppo, della lunghezza delle liste d'attesa e hanno proceduto a farla di tasca propria. Se il quadro era negativo prima della situazione pandemica, oggi lo è ancor di più. Come ben sappiamo, c'è da affrontare una carenza del personale sanitario e va fatto con assoluta urgenza. Il passo compiuto con l'emendamento che prevede la possibilità per i medici di famiglia e per i pediatri di andare in pensione a settantadue anni anziché a settanta è un primo passo. Bisogna certamente fare di più, ma la *ratio* della norma è contrastare la carenza di tutto il personale sanitario attraverso la valorizzazione di tutte le professionalità. Abbiamo approvato, inoltre, con questo decreto, la stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo assunto durante l'emergenza Covid. La misura riguarda coloro che abbiano maturato almeno diciotto mesi di servizio anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo che intercorre che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. Siamo riusciti a far diventare stabili questi lavoratori, che nel periodo della pandemia sono stati importanti, fondamentali, esponendosi tra l'altro in prima linea a contrastare il virus. modo, abbiamo voluto con forza inserire i 50 milioni del Piano oncologico nazionale, risorse stanziate che certo non risolveranno, ma contribuiranno a rispondere ai bisogni dei pazienti che devono avere la possibilità di essere di essere curati tempestivamente e nel migliore dei modi. Abbiamo prorogato di altri tre mesi lo *smart working* per le persone più fragili. L'Italia che guarda avanti è fatta anche, chiaramente, delle nostre fondamentali imprese. Penso alle attività commerciali e agli esercenti, ma più in generale alle attività economiche dei territori che hanno sofferto le restrizioni. Per questo motivo, tra l'altro, siamo intervenuti in materia di occupazione grazie sta facendo i conti con l'inflazione. Per questo in manovra abbiamo previsto importanti aiuti a famiglie e imprese. In questo decreto, nel settore delle costruzioni, abbiamo inserito la possibilità degli accordi quadro e dei prezziari per contrastare il cosiddetto caro materiali che sta creando serie difficoltà alle nostre aziende nella realizzazione dei lavori pubblici e nella conclusione dei cantieri con quelli del PNRR). Siamo intervenuti anche nel mondo dell'agricoltura, mi riferisco in modo particolare ai tempi per l'erogazione degli anticipi dei contributi alle imprese agricole, differendo al momento del saldo tutti gli adempimenti amministrativi, semplificando così le procedure e dunque cancellando tutta quella burocrazia che fa solo male al nostro Paese. L'agricoltura è e resta il centro della nostra azione politica, sosteniamo sempre chi lavora ogni giorno nella nostra terra. Siamo intervenuti sui balneari con una proroga di un anno delle concessioni: le spiagge per l'Italia sono un tesoro che non ha uguali, abbiamo il dovere di difendere un pezzo importante del tessuto socio-economico italiano, da Nord a Sud. Concludo con un passaggio sui Comuni. Nella nostra bellissima Italia ci sono tantissimi piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per questa realtà abbiamo previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per i segretari comunali, un sostegno economico ai piccoli Comuni che parte da quest'anno e terminerà al completamento del percorso del PNRR, quindi nel 2026. È un'attenzione importante che oggi viene confermata con un altro importante emendamento al milleproroghe per i Comuni fino a 5.000 abitanti, che estende la possibilità fino a ventiquattro mesi di mantenere la figura del segretario comunale titolare anche in altre sedi di fascia superiore. È una disposizione utile. L'emendamento approvato oggi è un passo in avanti soprattutto nell'ottica dell'attuazione, come dicevo prima, del PNRR, in cui i Comuni rivestono una parte fondamentale e sono in netta difficoltà nel raggiungere gli obiettivi e far sì che partano i cantieri. Certamente bisogna fare di più, è una battaglia - ne sono convinto - che non ha e non può avere colori politici, perché riguarda la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare Civici d'Italia-UDC-CI-MAIE, che sosterrà convintamente questo provvedimento.

Penso, ad esempio, al ragionamento che abbiamo fatto sul concorso svolto nel 2020, in cui chiedevamo di prorogare la graduatoria per

di fronte a migliaia di persone, che presentano i requisiti per essere messi in graduatoria perché hanno già passato i concorsi, si è detto di no.

nelle prefetture, nei posti in cui oggi siamo impegnati sul terreno per gestire la questione emergenziale. Non vorremmo avere in questo caso delle migrazioni particolari dettate dalla guerra che abbiamo in Europa.

dalla Commissione. Però, nello stesso tempo, nessuno può negare che siamo di fronte al fatto che abbiamo un rischio fallimento di migliaia e migliaia di

e 200.000 lavoratori rischiano di subire questo fallimento, perché da una parte si è voluto fare la guerra al superbonus, anziché correggerlo, e nello stesso tempo non si è risolto il problema dei crediti incagliati. Questo è il dato fondamentale. Cosa voglio dire, per concludere? Siamo di fronte al fatto che si è utilizzato il decreto milleproroghe per fare alcuni punti bandiera di propaganda elettorale, senza dare una risposta esaustiva e, nello stesso tempo, non si sono affrontati i problemi veri sulla precarietà, sul lavoro, sulle questioni che coinvolgono le persone dal punto di vista della loro esistenza. È per questo che noi convintamente votiamo un no secco alla conversione in legge di questo decreto-legge.

desideriamo innanzitutto ringraziare i presidenti della 1a Commissione Balboni e della 5a Commissione Calandrini per la conduzione dei lavori nelle Commissioni affari costituzionali e bilancio; conduzione avvenuta con grande equilibrio e senso delle istituzioni e delle prerogative dei parlamentari. Ancora una volta l'Aula del Senato si trova a esaminare e votare un decreto milleproroghe, uno strumento legislativo che dovrebbe servire come *extrema ratio* ed essere utilizzato in via eccezionale. Invece, in assenza di stabilizzazione normativa, occorre annualmente in soccorso per prorogare i termini di vigenza di disposizioni senza le quali si paralizzerebbero interi comparti pubblici e il funzionamento di settori essenziali per le imprese, i cittadini e i lavoratori. Si tratta di un provvedimento che, in un ordinamento maturo e completo, non dovrebbe esistere, ma che evidentemente è figlio dell'incapacità dell'incapacità dei Governi di dare stabilità a norme importanti in tutti i settori vitali del Paese, dalla sanità alla giustizia, dalla scuola all'industria e al sociale. La seconda osservazione è di carattere politico e riguarda l'avvenuta proroga, da parte di questa nuova maggioranza, di molte misure già in essere e, come tali, pensate e volute dai Governi precedenti, Governi ai quali Fratelli d'Italia si era in passato fieramente opposta fuori e dentro il Parlamento, ma che oggi evidentemente apprezza, almeno in alcune parti, mostrando in tal modo la chiara incoerenza della propria azione propagandistica. Mi riferisco alle norme sul 4.0, con la proroga a novembre del termine di consegna dei macchinari per le imprese che vogliono investire utilizzando i relativi crediti di imposta, e alla proroga dei termini per mettere a terra tutte le norme del *family act*. Penso alla conferma dello *smart working* per i lavoratori fragili; penso ai fondi per Radio Radicale e per il settore editoriale e alla proroga dei prezzari nell'ambito degli accordi quadro dei lavori pubblici.

ma che vede invece confermati solo i passi avanti decisi da altri: la proroga della ricetta elettronica al 2024; la proroga dell'incarico ai medici specializzandi per supplire alla carenza di personale medico; la proroga per l'utilizzo del fondo per la riduzione delle liste d'attesa; la proroga per la stabilizzazione del personale sanitario amministrativo precario che ha lavorato durante la pandemia. La terza evidenza riguarda l'utilizzo strumentale, finanche dannoso per l'Italia, del provvedimento proroga termini. Lascia inoltre disorientati la disapplicazione a piacere della normativa sulla concorrenza: no per il balneari; sì invece per un settore vitale, ancora più in un periodo di grave crisi energetica, come quello delle grandi concessioni di derivazione idroelettrica. Dietro questo incongruenze non c'è una visione strategica, ma solo il chiaro intento di rispondere a interessi particolari. Nemmeno nel contrasto al rischio idrogeologico si fanno passi avanti. Brillava il recente impegno del Governo, con l'ordine del giorno approvato, a ripristinare la cabina di regia, proseguendo così un vero lavoro strutturale che eviti ai territori di franare, ai fiumi di esondare e alle persone di morire. Lì ci limita solo a prorogare misure in essere, come la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, tamponando l'emergenza fino al 31 dicembre 2024. Apprezziamo naturalmente, come Gruppo Per le Autonomie, l'attenzione che è stata dedicata ad alcune delle nostre proposte. Mi riferisco in particolare alla proroga per l'utilizzo della compensazione del credito d'imposta sul carburante agricolo: una boccata d'ossigeno per le aziende agricole italiane, colpite dall'esplosione dei costi dell'energia; riferisco alla proroga al 31 dicembre 2023 del termine per le modifiche statutarie degli enti del terzo settore, necessarie per l'iscrizione al nuovo registro unico nazionale del terzo settore;

che ci ricordano quanto l'Italia in tutti questi settori sia invece in attesa di interventi definitivi e delle riforme strutturali previste dal PNRR. Il provvedimento in esame, pesantemente corretto da emendamenti parlamentari, anche della stessa maggioranza, verrà convertito di fatto con il solo esame del Senato, con il metodo quindi del monocameralismo alternato. Nonostante siano passati diversi mesi, sulle questioni economiche Governo e maggioranza non hanno ancora definito una precisa strategia. di conoscere come si intenda sostenere la crescita; come si intenda favorire la competitività del sistema produttivo; come si vogliano difendere cittadini e imprese dal caro energia, da aprile in poi; e anche come si intenda in generale difendere il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni. Tutte domande che, purtroppo, non hanno ancora ottenuto una risposta compiuta.

una differenziazione su tre qualificazioni di questo decreto, analizzando dapprima il metodo, poi il merito e poi lo scenario dentro il quale questo provvedimento si muove e rispetto al quale avrebbe dovuto dare risposte, a mio avviso, più convincenti. Prima il metodo:

di recepire le istanze dell'opposizione e, come mi pare dicesse prima il collega Patton, anche un atteggiamento istituzionalmente molto corretto. Voglio riconoscerlo, perché penso che, quando lavora bene il Parlamento e quando c'è rispetto delle varie componenti politiche e dei vari Gruppi, ci sia anche un lavoro prezioso per la democrazia. Allo stesso modo, voglio riconoscere l'atteggiamento positivo del ministro Ciriani

ci ha seguito e che è stata sempre presente ai lavori della Commissione. Questo ve lo dovevo, perché a me non piace non riconoscere anche agli avversari i loro meriti. Con la stessa nettezza, però, vi voglio anche dire che, dal punto di vista del merito,

Come abbiamo fatto anche con l'avvio di questo Governo, abbiamo cercato di tenere un atteggiamento il più possibile propositivo (dirò

Facciamo un esempio. Avete lavorato sul tema della proroga dei medici, e io credo che fosse una misura inevitabile, però restano provvedimenti tampone. Come si fa a non partire dal dato - rivelato oggi dal ministro Schillaci - dei 10.000 esodi immediati che hanno la necessità di un intervento strutturato, radicale dal punto di vista della sua organicità, sul tema delle liste d'attesa, sul tema dei pronto soccorso e su quanto è necessario per non far collassare il sistema. State molto attenti, e lo dico non perché auspico questa cosa, ma se c'è un tema di emergenza sociale in questo Paese non è il reddito di cittadinanza: è il collasso sistematico della sanità, che rischia di venire addosso a tutti noi. quindi aspettata una visione o in legge di bilancio o in questo provvedimento, e non l'ho trovata. Continuate a parlare di autonomia differenziata sulla questione della sanità. Penso che dovremmo avere

dal 31 marzo al 31 maggio gli interventi del PNRR sul tema di edifici scolastici, asili e scuole d'infanzia; le

ho l'obbligo di darvi un ammonimento, un avvertimento: quel codice non semplifica alcunché, contiene 230 articoli; è il codice delle complicazioni, non delle semplificazioni.

la nostra forza politica, il terzo polo, ha elaborato, per avere qualche risposta convincente su questo punto. Così, però, mettete a rischio il PNRR; quindi, è inutile che proroghiate le norme sugli asili, quando non riuscirete a fare le gare per migliorare la vita delle donne, la libertà delle famiglie e i principi educativi per i ragazzini.

avete prorogato almeno in quota parte Industria 4.0, avete eliminato Formazione 4.0, e chiaramente la cosa ha un rilievo e una pesantezza. Penso che tutto questo, insieme alle proroghe ad esempio per i medici a settantadue anni, sia inevitabile, perché è inevitabile in questo momento avere qualche medico in più sul campo.

delle quali avete discusso. Non vi siete interessati di discutere di qualcosa in più rispetto a Industria 4.0 o di qualcosa di meglio sul tema della sanità. No,

perché sapete perfettamente - e lo spettacolo dato oggi lo conferma - che quell'iniziativa porterà a una conseguenza grave sul piano europeo; che non si tratta di una vera proroga; e che non aiuterete a salvaguardare gli investimenti di chi ha investito. È invece del tutto evidente che, se in questo Paese arriverà un giovane, magari talentuoso, magari con un'idea diversa, capace di competere anche sulle iniziative sul litorale di carattere culturale e turistico, quel giovane non avrà nessuna possibilità, perché le *lobby* avranno sempre la meglio.

dubbio. Diciamoci la verità, avete creato le condizioni per uno schema molto, molto debole. Meno male - e lo dico con un atteggiamento non privo di orgoglio il terzo polo ha continuato un atteggiamento positivo e propositivo nei vostri confronti. Che cosa abbiamo fatto? In conclusione, abbiamo portato avanti il tema della proroga al 2023 a proposito degli operatori delle professioni sanitarie,

di scrivere i decreti attuativi sul *family act*, dando conseguenza a quella grande iniziativa voluta dalla nostra ministra Bonetti. Abbiamo fatto in modo che ci fosse un adeguamento sui prezzari dei lavori pubblici. Abbiamo attuato o avuto soddisfazione su una proroga di Industria 4.0. Abbiamo chiesto più mesi per la riforma delle fonti energetiche. Abbiamo messo qualche risorsa in più su Radio radicale.

interviste e dichiarazioni di Ministri che si sono avvicendati e che avevano promesso di chiedere un maggior controllo nel Ministero delle infrastrutture dei trasporti sugli investimenti dei concessionari autostradali, che - lo ricordo a tutti - non sono i padroni di quel bene, ma lo gestiscono provvisoriamente.

iniziativa tesa rafforzare il ruolo del Ministero è andata avanti, nessuna richiesta puntuale sul tema degli investimenti è stata operata. Ho presentato un emendamento, con che ogni anno i concessionari autostradali consegnino al Ministero e al Parlamento la relazione puntuale dei loro investimenti sulla nostra rete.

Siamo al terzo minuto, senatrice Paita. PAITA *(Az-IV-RE)*. Non ci siamo arresi e sono veramente felice di dire che tutte le forze politiche alla fine questa iniziativa l'hanno sostenuta. Cambierà qualcosa, avremo delle reti più sicure? Sicuramente saremo più in grado di controllare. Spetterà a noi questo compito gravoso e impegnativo. Volevo chiudere con una battuta finale: potevamo con questo provvedimento fare cose davvero impegnative e forti per il Paese. Avete scelto la logica del massimo ribasso, vi siete concentrati su battaglie ideologiche che non porteranno nulla agli italiani e per questa ragione non potremo votare a favore, ma con la stessa lealtà vi diciamo che, se se ci sarà su questi temi un'iniziativa più forte nei prossimi mesi, sicuramente valuteremo di volta in volta i singoli provvedimenti, pensiamo che, soprattutto in provvedimenti come il milleproroghe, l'atteggiamento ideologico non porti a nulla. Certamente però, di fronte a un impianto così fragile e di così poco respiro, il nostro voto non può che essere contrario.

Voglio partire dai temi che in parte modificheranno il mio intervento, perché la senatrice Paita ha detto cose in alcuni casi molto condivisibili, però con troppe dimenticanze. La prima, condivisibile in assoluto, è che anche noi crediamo che si sia fatto davvero un buon lavoro: il Senato ha fatto ciò che doveva fare.

come dovrebbe sempre fare, ha fatto un lavoro di arricchimento: questo è il lavoro del Parlamento. Anche in questo mi sento di condividere le valutazioni dei colleghi che prima di me hanno voluto sottolineare la positività di questo comportamento e di questo provvedimento, soprattutto perché - com'è giusto che sia e così è stato - molti degli emendamenti sono stati approvati senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Non ho contato se fossero più quelli di maggioranza o di opposizione, ma davvero si è guardato al merito e si è dato risposta alle istanze che venivano poste.

Innanzitutto, sul tema sanitario, sul quale tornerò in seguito, sia con l'emendamento Ronzulli, sia con l'emendamento Ternullo, si sono date risposte importanti al nostro Servizio sanitario nazionale, ma è evidente che non poteva essere questo il provvedimento e il luogo in cui andare a risolvere i problemi della sanità nazionale o regionale; non poteva essere questo il provvedimento, così come non poteva essere una legge di bilancio, che - non possiamo dimenticarlo - è stata approntata e portata ad approvazione da parte di questo Governo in quindici-venti giorni di tempo. È evidente che si è adottato uno schema che veniva dal precedente Governo. Arriverà il momento in cui si metterà mano e lo dico perché sono d'accordo, a partire ad esempio dal fatto che probabilmente - lo penso io, ma lo pensano in molti - il numero chiuso a medicina non ha più motivo di essere e dev'essere superato.

nostro Paese. Non devo essere io a difendere il ministro Salvini, ma la collega senatrice Paita, visto il ruolo che ricopriva nell'altro ramo del Parlamento, sa bene che questo codice degli appalti ci arriva dall'allora ministro Giovannini non è stato approntato dall'attuale Governo. I tempi del PNRR portavano alla presentazione del codice degli appalti entro il 31 dicembre 2022, dunque è stato portato dal ministro Salvini, ma è evidente che il lavoro è stato fatto in particolare dal sottosegretario Bellanova,

contro il parere del precedente Governo, che - come ricorderà - avrebbe voluto addirittura che non tornasse alle Camere per il parere. Invece è tornato, grazie a un emendamento che la Commissione di cui ero membro ha chiesto ed approvato

Anche chiudendo il codice degli appalti così come ci è arrivato, sicuramente non si risolve il problema, ma ci saranno ancora cose da affrontare.

a colmare lacune, a risolvere situazioni e a dare più respiro ad altri provvedimenti che non hanno avuto possibilità di averne a sufficienza. Il tutto affinché ci sia uno spazio adeguato

senatrice Ronzulli, che consente agli operatori delle professioni sanitarie, infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione di operare in regime privato, *extra moenia*, in un momento delicato come questo, che è ancora definito come post-Covid, per un monte ore settimanale raddoppiato, non superiore alle otto ore, fino al 2023, quando la normativa prevedeva quattro ore settimanali, fino alla fine dello stato di emergenza: anche questo è dare risposte. consente poi il reclutamento del personale medico e infermieristico straniero, in deroga. La situazione è questa, lo sappiamo e lo vediamo: anni di numero chiuso a medicina non hanno prodotto le risposte che invece oggi il Paese chiede. quindi possibile, grazie ad un emendamento, operare in Italia in regime di equipollenza di titoli, fino al 2025, in deroga alle norme di riconoscimento della professione. Finora era consentito fino alla fine del 2023 e noi lo portiamo al 2025, per avere respiro e dare la possibilità

stesso vale per l'emendamento della collega Ternullo, che proroga la stabilizzazione del personale sanitario, per rafforzare il sistema sanitario, fronteggiando anche in questo caso la grave carenza di personale. Dopodiché, cito un emendamento trasformato in ordine del giorno: ci accontentiamo, ma

31 dicembre 2024 rispetto al 2023, togliendo il limite del 30 giugno 2023 entro cui si doveva effettuare il 60 per cento dei lavori. Pertanto, ampliando la possibilità di risposta sul tema dell'edilizia economico-popolare, credo si faccia davvero una grande

è un tema che riguarda il nostro Paese, che ha le coste più lunghe d'Europa e si ritrova - guarda caso - ad essere esposto alla direttiva Bolkestein, anche due o tre anni fa lo stesso Bolkestein, venendo a Roma, ha detto chiaramente che la propria direttiva non poteva e non doveva essere applicata in questo contesto. È accaduto proprio questo e facciamo finta di nulla. Vorrei inoltre capire perché la Spagna è esonerata da tutto ciò, perché le sue coste rimangono agli spagnoli, mentre noi dobbiamo esporci agli appetiti, in particolare dei tedeschi, ma non solo, che evidentemente, non avendo il mare, vedono nelle nostre coste una ghiotta occasione anche per portare i propri

non parliamo però di situazioni in cui spesso ci sono aziende familiari che da tempo lavorano sul territorio, dando risposte che assicurano un'accoglienza familiare ai turisti italiani e stranieri che vengono in Italia.

i cittadini italiani che andranno a prendere un ombrellone pagheranno di meno, credo che sia sulla strada sbagliata, che non sia su quella giusta. Dopodiché, se c'è da rivedere le tariffe, lo si faccia; si proceda a una mappatura per capire davvero com'è la situazione italiana; però, se la mappatura è in ritardo (come lo è),

che esaminiamo oggi mostra tutte le contraddizioni delle facili promesse elettorali e rappresenta un'altra occasione mancata per questo Governo, ma soprattutto per il nostro Paese. La finzione infinita della ricerca di una direzione coerente si trasforma in una serie imbarazzante di convulsioni, di retromarce e di giravolte giravolte delle forze politiche di maggioranza che sostengono questo Governo, contraddizioni che abbiamo anche riscontrato nello stesso partito di cui il Presidente del Consiglio fa parte. La schizofrenia di questo Governo colpisce in maniera catastrofica in primo luogo il superbonus. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti, anche quelli di altre forze politiche, che abbiamo voluto presentare proprio per impedire la catastrofe. Ma ecco la contraddizione a cui accennavo prima: anche Fratelli d'Italia e Forza Italia presentano e segnalano emendamenti per prorogare il superbonus. Mi sono chiesta e se lo sono chiesto anche le molte imprese che avevano sperato in un cambio di rotta di questo Governo. Io l'ho trovata, una risposta, colleghi: secondo me volevano metterci una pezza, metterci una pezza, perché smantellare il superbonus e non affrontare la questione della cedibilità dei crediti è un imperdonabile autogol, sì, del Governo, ma anche delle forze politiche che lo sostengono. *(Applausi)*. 90.000 cantieri bloccati e migliaia di imprese sull'orlo sull'orlo del fallimento: una situazione insostenibile, che in altri Paesi basterebbe a far dimettere un Governo. Se la domanda è eccessiva, il fatto di togliere il reddito di cittadinanza e il lavoro a milioni di imprese certamente la farà contrarre. Queste le convinzioni del Governo in carica. Quale altro motivo può esserci per distruggere 900.000 posti di lavoro? Ma lotteremo contro questa schizofrenia e contro questo cinismo. Noi del MoVimento 5 Stelle nelle Regioni e in Parlamento interverremo sempre per sbloccare i crediti e agevolare incentivi che hanno migliorato il conto dell'Italia sul PIL nel 2021 e nel 2022, sul lavoro e sul taglio delle emissioni inquinanti. È solo questo il motivo alla base dei nostri emendamenti e dell'ordine del giorno. Colleghi, non si abbatte l'inflazione togliendo dignità e lavoro ed eccola, dunque, la coerenza nascosta dai proclami: non ci si poteva aspettare nulla di diverso da un Governo di destra-centro, come amate definirvi. Per mesi, il grido d'allarme delle 90.000 imprese è stato ignorato da un Governo di chiara ideologia di destra, la stessa ideologia che consente di non ridurre le accise e l'IVA sui prodotti energetici, la stessa ideologia che non proroga il reddito di cittadinanza e la stessa ideologia che ripropone la lotta di classe nella forma più estesa possibile, facendo la guerra senza quartiere ai poveri, alla scuola, alla sanità e al Sud. La presidente Meloni ha dichiarato che il reddito di cittadinanza va tolto, perché ha fallito tutti i suoi obiettivi. Mi chiedo, colleghi, e lo chiedo anche a voi: ma prima di spingersi in quest'affermazione, la presidente Meloni ha cercato il confronto con il territorio? Possibile Possibile mai che un Governo attui in pochi mesi un provvedimento così importante solo perché a certi caporali mancano le braccia a 1,5 euro l'ora? Lo chiedo con il cuore, oggi, a voi del Governo e a voi colleghi: confrontatevi con i sindaci, chiedetelo a loro se questa misura economica non è riuscita a sollevare i Comuni dall'impotenza di non poter dare una mano a chi ne ha bisogno. Chiedetelo agli assistenti sociali e ai volontari che lavorano nei territori se il reddito non rappresenti uno strumento fondamentale di protezione sociale. Confrontatevi con i prefetti, con le Forze dell'ordine. Io l'ho fatto, forse perché vivo in una città complessa, ma anche molti di voi qui presenti vivono in aree complesse. C'è un rischio concreto che la mancanza di misure di protezione economica porti porti a un inevitabile effetto incrementale dei reati e non solo di quelli di poco conto. È nota a tutti noi la grande capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali dove lo Stato arretra e non funzionano le inutili ciarle che raccontano che i poveri starebbero ricattando lo Stato, meno reati in cambio del reddito. Colleghi, gli occupabili sono una categoria inventata, come se chi è disoccupato lo fosse per scelta. Eliminati i *navigator*, origine di tutti i mali d'Italia, quali investimenti sono stati fatti per implementare le politiche attive del lavoro? Tra qualche mese toglieremo il reddito di cittadinanza a migliaia di padri di famiglia. Bene, dove sono i corsi obbligatori di formazione e di

Proprio quel Governo di destra-centro ha indetto l'avviso per 1.200 funzionari da impiegare nei centri per l'impiego, e per la Sicilia 1.200 posti di lavoro in più non sono pochi, solo a fine dicembre 2021 e ancora non abbiamo gli esiti. Mi sono fatta anche un'altra domanda, che pongo anche a voi, colleghi. Come si può conciliare quanto detto sinora con la risoluzione sul reddito minimo presentata dal Consiglio d'Europa *(Applausi)* che la ministra Calderone ha approvato? In Italia lo abolite, ma lo votate in Europa. Cos'è, schizofrenia? Disturbo bipolare? Per me è certificazione della malafede, imposta dal vostro rapporto poco facile e poco felice con l'Europa. Si vede proprio nei tre emendamenti riformulati sulla questione delle concessioni demaniali, che ci porta a uno scontro con Bruxelles, che con ogni probabilità probabilità ci porterà a una procedura d'infrazione, come quella ricevuta dal Portogallo da parte della Commissione europea, senza neanche risolvere il problema alle imprese, perché le abbiamo mantenute nell'incertezza. Stessa identica cosa con la direttiva casa *green*, che il Governo e poi contesta, alimentando paura senza però trovarvi soluzioni. Come il MoVimento 5 Stelle ha chiaramente indicato nel suo programma elettorale, serve con urgenza un piano industriale sulla casa, basato sulla stabilizzazione

chiedendo la proroga di almeno sei mesi per definire e portare a gara tutti i progetti inseriti nel fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, proroga che, tra l'altro, ha ottenuto un parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni, che voi però vi ostinate a non concordare. Intere opere necessarie, a cui manca veramente poco per essere realizzate, che sono state frutto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, che non hanno personale a disposizione, dovranno attendere e fermarsi in attesa della vostra ricognizione e dell'approvazione dei piani di sviluppo e coesione che ad oggi non ci sono e non per colpa degli enti locali, ma del Ministero competente. Mi chiedo allora, e lo chiedo anche voi, colleghi, come faranno i Comuni a fermarsi o a continuare l'*iter*, se non c'è ad oggi la possibilità giuridica di trasferire Stiamo chiedendo ai Comuni di fermarsi. Mettiamo il caso che questa riprogrammazione avvenga nel più breve periodo, come mi auguro, e che tutti i progetti automaticamente passino nei piani 2021-2027, cosa succederà

ambiti territoriali; sono nati per il Sud, per quei paesi che devono superare dei *gap*. La riprogrammazione delle somme non spese non può rappresentare l'ennesimo scippo ai cittadini di quei territori. Per concludere, vorrei già dare la comunicazione che, per tutte le motivazioni che ho elencato, nonostante molti emendamenti da noi presentati siano stati accolti dal Governo, lo strumento, l'atto normativo presentato era privo di notevoli argomenti e temi che devono essere affrontati. In Commissione abbiamo lavorato duramente ed è per questo che ringrazio davvero per la professionalità dimostrata e il lavoro immane svolto dai Presidenti della 1a e della 5a Commissione, che hanno hanno diretto i lavori in maniera veramente ottimale e quasi al di fuori di ogni aspettativa; di questo li ringrazio. Ma purtroppo l'atto, così come è scritto, non può che avere il voto contrario da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Questo ringraziamento ai Presidenti non è di prammatica, ma segnala un qualcosa di più importante e profondo: segnala un ritorno della democrazia parlamentare. *(Applausi)*.

indice di un impatto sicuro del Parlamento sul provvedimento e di un impatto senza particolari preclusioni di parte o di ruolo. C'è stato un momento che vale vale la pena ricordare, perché i lavori in Commissione spesso non sono noti all'esterno. Credo che i Resoconti vengano letti veramente da poche persone; ma ricordo a tutti che, volendo, possono leggerli e capire come si arriva a questi provvedimenti. C'è stato un momento in cui alcuni emendamenti del Governo sembravano sovrapporsi agli emendamenti presentati dagli onorevoli senatori. c'è stata una franca discussione all'interno della Commissione e si è deciso che invece la primazia dovesse essere mantenuta sugli emendamenti presentati dai senatori.

con il giusto aspetto di avvocato del Parlamento. Siamo passati dal sedicente avvocato del popolo italiano all'avvocato del Parlamento,

(che nessuno sa cosa sia, io ho guardato tante volte la Costituzione e ho continuato a leggerla, cercando cosa diamine fosse questa cabina di regia, ma non l'ho mai trovata) voto di fiducia. Questa era la trafila. Così facendo è un po' meglio e speriamo di riuscire ad arrivare al completamento della democrazia parlamentare, che è quello della seconda lettura.

Perché dopo dieci anni, in nove dei quali ha governato la sinistra, quello che ci rimane è un Paese che va avanti a continue proroghe, con un continuo portare avanti, un continuo mettere la sabbia sotto il tappeto e sperare che qualcun altro la pulisca. A tal proposito, porto un esempio paradigmatico. Io ho potuto solo ascoltare l'intervento della collega Damante del MoVimento 5 Stelle con un sopracciglio alzato, perché sembra che il superbonus sia colpa nostra.

della scorsa legislatura fosse il MoVimento 5 Stelle. E non capisco perché non abbiano ancora sistemato la questione del superbonus, quando avevano tutto il tempo per poterlo fare; tutta la forza parlamentare poteva farlo. *(Applausi)*. Io ricordo, però, che all'epoca, nella scorsa legislatura, quando arrivavano i comitati e i rappresentanti delle imprese a chiedere rispondevano fischiettando: sì, chissà, vedremo. Ecco, passata una legislatura a fischiettare, non si fa in tempo a tornare all'opposizione ed eccoli subito trasformati in leoni. Bisogna sistemare tutto! No, non si può sistemare tutto, perché, nel disastro che hanno fatto sul superbonus, i cocci sono talmente tanti che è impossibile impossibile raccoglierli tutti e si cerca di fare il possibile. Comunque, in ogni caso, ripeto che il tempo per sistemare il superbonus, tutti i modi e tutti i voti li avevano nella scorsa legislatura. Questo Paese precario, questo Paese a scadenza è un danno per le nostre imprese; è un motivo della nostra scarsa crescita e della impossibilità di raggiungere altre economie, che in questo momento si sono già riprese dai massimi pre-pandemia e pre-crisi, mentre noi siamo largamente arretrati rispetto a quei livelli. Ma questo è ovvio: se si sta parlando di orizzonti temporali molto brevi e continuamente prorogati, senza nessuna certezza che queste proroghe vadano in porto, chi mai investe? Chi mai riuscirà a fare una programmazione a lungo termine, laddove, quando l'imprenditore mette soldi, deve essere sicuro di poter portare a termine quello che i suoi investimenti stanno iniziando? E la questione dei balneari non è estranea a questo ragionamento.

quale imprenditore può andare a mettersi in una situazione del genere? E questo perché? Per delle direttive europee che arrivano da Paesi senza il mare! Qui siamo sempre nello stesso capitolo di alcuni provvedimenti su cui noi stiamo preparando battaglia, quale quello sulla casa *green*. Perché qui si prevedono investimenti sulle case che tengono bene dentro il calore? Ma secondo voi, in Sicilia, in Calabria, Calabria, in Campania, il problema è fare una casa che tenga bene dentro il caldo o una casa antisismica, tanto per dire? Secondo me, sarebbe meglio fare una casa antisismica, il problema è che chi decide in questo momento in Europa è un Paese dove fa molto freddo e non ci sono i terremoti. Quindi, guarda caso, arrivano queste misure. Oltretutto, in quei Paesi non ci sono i borghi medievali che caratterizzano il nostro Paese. E noi dobbiamo difendere le specificità del nostro territorio. Non dobbiamo andare dietro a direttive che, in certi casi, sono totalmente sbagliate. Vorrei aggiungere alcuni punti che siamo riusciti, con il lavoro parlamentare e con gli emendamenti,

sarà importante la manutenzione dei ponti del bacino del Po? Eppure, poiché devono esserci delle scadenze per i contratti, si rischiava di lasciare svanire

e l'accademia di Imola. Vogliamo dire che sono un tesoro per il nostro patrimonio formativo, che vengono da tutto il mondo per studiare in Italia, e che quindi sono una ricchezza per il nostro Paese oppure le consideriamo ogni volta questioni che devono essere finanziate di volte in volta, col cappello in mano, come se ci fosse bisogno di un'elemosina? Ecco, sarebbe opportuno - lo sogno - un Paese

è stata fondamentale per una stagione indimenticabile del nostro turismo, abbia i fondi per poter rinnovare la flotta; dovrebbe essere considerato un investimento e un patrimonio di tutti, perché porta utile, porta turismo e PIL, che ci consente di

un auspicio rispetto a questo milleproroghe è che sia uno degli ultimi; che tutti i prossimi provvedimenti siano stabili e definitivi, in modo tale da poter dare certezze ai nostri imprenditori e ai nostri lavoratori. Il nostro voto sarà ovviamente a favore di questo provvedimento. Presidente, ministro Ciriani, colleghi e colleghe, il provvedimento cosiddetto milleproroghe, ha sempre rappresentato, a mio avviso, un'occasione importante per ampliare misure utili al Paese: per le famiglie, le imprese, gli enti locali, l'istruzione, la salute, il lavoro. L'auspicio del collega Borghi è molto ambizioso, perché il proroga termini ha sempre seguito la legge di bilancio. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un vuoto: nelle politiche economiche e sociali non siamo in presenza di una corretta programmazione economica e sociale. Penso alla legge di bilancio, per il poco tempo e anche, secondo me, per una scelta che riteniamo sbagliata da parte della maggioranza: quella di non centrare gli obiettivi reali del Paese, di non comprendere che oggi la priorità deve portarli a riflettere sulle questioni sociali aperte, sulle disuguaglianze che si ampliano per effetto di salari incompatibili con la qualità della vita delle persone. dunque in presenza di un proroga termini senza un'identità perché manca l'identità della legge di bilancio e mancano le programmazioni e le priorità da parte di questa maggioranza rispetto alle questioni economiche e sociali, che, per un Governo politico, dovrebbero rappresentare il cuore della propria iniziativa. Non condivido il trionfalismo della maggioranza rispetto ai primi cento giorni; lo voglio dire con grande chiarezza, perché se i loro risultati consistono consistono esclusivamente nei risultati elettorali ottenuti anche la settimana scorsa nelle elezioni nel Lazio e in Lombardia, io continuo a pensare, invece, che questi primi cento giorni abbiano mostrato un vuoto terrificante proprio sulla capacità di questa maggioranza di leggere le questioni sociali ed economiche in atto in questo Paese. *(Applausi)*. Colleghi, la prima cosa da fare è restituire al lavoro la priorità che il lavoro merita; correggere le enormi disuguaglianze in atto in questa società, in questa comunità, in questo Paese, che spingono sempre di più verso forme di solitudine e di povertà un numero sempre più elevato di persone. Voi avete fatto il contrario: anziché occuparvi delle dinamiche sociali, avete scelto forse la strada più semplice, quella della propaganda (lo capisco), quella di discutere per settimane e settimane del tetto sui contanti, quella della demolizione degli strumenti elettronici

sulla proroga termini abbiamo assistito a tante forzature, come gli interventi del Governo per sopprimere emendamenti dello stesso Governo che aveva riformulato emendamenti del Parlamento. Sono forzature che mostrano tanta confusione e, soprattutto, una difficoltà ad intraprendere la strada delle priorità. Questo è un punto politico per noi fondamentale, dal quale vogliamo partire. Lo dico con chiarezza: abbiamo riconosciuto - e lo voglio fare anch'io in Aula - al ministro Ciriani e al presidente Calandrini, ai relatori senatori Balboni e Damiani il fatto di aver definito un percorso corretto di analisi degli emendamenti in Commissione. Questo ha restituito sicuramente un po' di centralità al Parlamento; ha ribadito che si possono avere idee diverse, ma che su alcune questioni si possono anche intraprendere strade condivise nell'approvazione di numerosi emendamenti. Noi non discutiamo la questione di metodo, che continuo a pensare che oggi sia stata positiva grazie alla disponibilità del Ministro e anche dei Presidenti delle due Commissioni. Quello che non c'è in questo decreto-legge è l'identità, la priorità, quegli elementi fondamentali di proroga che sarebbero stati indispensabili e necessari. Voglio partire anche dalla correzione che avevamo proposto e che intendo qui sottolineare, perché per noi è una questione cruciale. Avremmo preferito che aveste ammesso da subito l'errore fatto, durante la legge di bilancio, di modificare opzione donna, perché lì sì che avreste aiutato 20.000 donne ad evitare di rimanere nella solitudine e nella precarietà. Avremmo preferito un intervento ancora più rilevante sulle dinamiche sociali del lavoro fragile. Certo, anche grazie alla nostra caparbia determinazione di svolgere un ruolo propositivo e di opposizione, all'ultimo - devo riconoscerlo al Governo -, dopo aver bocciato un nostro emendamento, avete introdotto un emendamento riformulando anche il nostro che era stato respinto. Questo significa quindi che fare opposizione serve. Lo dico innanzitutto ai colleghi di Fratelli d'Italia: provate ad abbandonare questa litania costante nel fare opposizione al passato. Gli elettori vi hanno consegnato legittimamente una responsabilità di Governo. Se continuate a perdere tempo sul passato, dimenticate per intero i problemi del presente e, soprattutto, non individuate il futuro corretto per questo Paese. Lo dico con grande franchezza e chiarezza tra di noi: questa litania ormai è priva anche di fondamento, perché i due terzi delle componenti di questa maggioranza di Governo hanno governato nell'ultima legislatura; una componente ha governato per un intero anno della legislatura e l'altra componente ha governato, negli ultimi vent'anni, per oltre dieci anni. Quindi anche questa litania sulla contrapposizione al passato non è coerente nemmeno con la composizione di questa maggioranza, ed è per questa confusione che si determina una mancanza di obiettivi da parte di questa maggioranza e continua ad esserci tanta confusione. Avremmo preferito poter affrontare da subito il tema della sanità. Avremmo preferito che si fosse ammesso il problema fondamentale, perché la sanità è un diritto universale in questo Paese e senza le risorse necessarie, senza un ritorno almeno a una quota del 7 per cento del PIL, non riuscirete a chiudere i bilanci delle Regioni, lasciando la sanità pubblica nel caos, rendendo non esigibile il diritto universale alla salute. Avremmo preferito che si fosse deciso di lavorare anche sui vostri manifesti elettorali, poi negati quando vi siete trovati di fronte alla responsabilità di Governo. Avremmo preferito le proroghe sulle accise, per aiutare tante famiglie ad evitare un caro del costo del carburante insostenibile ed iniquo *(Applausi)*, perché picchia in maniera disomogenea, come tutto il sistema dell'inflazione,

noi ampliamo le disuguaglianze, spingiamo nella solitudine, nell'indifferenza e nella povertà un numero sempre crescente di famiglie italiane. Avremmo preferito che si fossero prorogate le misure agevolata al 5 per cento sul metano da autotrazione, perché lì avremmo dato un vantaggio anche a coloro che hanno investito per migliorare le emissioni in atmosfera, per ridurre le fonti di inquinamento, sia nell'autotrasporto privato, sia nel sistema del trasporto delle merci, dove sono stati fatti investimenti da tantissime imprese che oggi si vedono un costo del metano insostenibile per la capacità di stare sul mercato. Avremmo preferito che non lasciaste nella solitudine anche la rete della distribuzione del metano per autotrazione, che a proposito di idrogeno potrebbe rappresentare un veicolo essenziale per impostare un'innovazione straordinaria in questo Paese. Paese. Vi abbiamo chiesto proroghe significative sull'energia, che invece sono state marginalizzate, derubricate e respinte. Allora, questo è il problema, onorevoli colleghi: c'è molta confusione, come sui balneari, e assistiamo anche ad un pericoloso rigurgito antieuropeo che io definisco a targhe alterne, perché la vicenda dei balneari è significativa. Avevamo chiesto da subito un comportamento coerente e trasparente del Governo per avere una relazione tecnica, corredata dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, che certificasse l'assenza di oneri sulla finanza pubblica. Non avete fatto un intervento utile alle imprese; anzi, potevate fare un intervento utile alle imprese italiane, ma avete reso più precaria l'impresa balneare, quella legale, quella che investe, quella che chiede futuro e garanzie per poter realizzare gli investimenti. Voi avete utilizzato Eurostat (a proposito di rigurgiti antieuropei a targhe alterne) per non affrontare il tema della cessione dei crediti sul superbonus, dove spingete decine di migliaia di imprese verso procedure fallimentari per mancanza di liquidità; avete cioè rinunciato ad affrontare le priorità, ancora continuando sulla propaganda. Credo che sia giunto il momento di cambiare rotta, di rivedere le priorità nelle politiche economiche e vedrete che sarà meno difficoltoso un proroga-termini coerente con i bisogni reali del Paese e con i bisogni reali delle imprese e delle famiglie italiane.

anche a tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione delle Commissioni 1a e 5a riunite. Ringrazio veramente di cuore anche per gli attestati di stima che sono arrivati, in modo trasversale, da tutti i componenti non solo della Commissione, ma anche

grazie alla sua capacità e alla sua ostinazione nel rimettere al centro le Aule parlamentari e le aule delle nostre Commissioni. Condivido anche ciò che ha detto prima di me il collega senatore ha dichiarato che abbiamo fatto un buon lavoro in questo decreto milleproroghe. Aggiungo che lo abbiamo fatto per l'Italia e dobbiamo essere orgogliosi di questo, perché abbiamo dato un segnale molto forte di serietà,

in questo lavoro e lo voglio ribadire perché è molto importante questo metodo che abbiamo condiviso, che potrà tornarci utile anche per il futuro, quando tra qualche mese inizieremo a lavorare sulla legge di bilancio. Abbiamo svolto 50 audizioni, abbiamo definito 360 emendamenti segnalati abbiamo incassato le istruttorie dal MEF, cosa che negli anni passati - posso garantirlo agli amici e ai colleghi che non c'erano nella scorsa legislatura - non è mai accaduta. I grandi problemi che abbiamo avuto, in passato, derivavano dal fatto che non arrivavano i pareri e le istruttorie da parte del MEF.

Vorrei anche ricordare una cosa molto importante, in particolare al collega senatore Manca, a cui ho sentito fare riferimenti non molto condivisibili, dicendo che abbiamo che abbiamo scelto la propaganda, che abbiamo fatto molte forzature e che non condivide l'ottimismo per i primi cento giorni di Governo. Io invece dirò il perché condivido l'ottimismo per i primi cento giorni di Governo. Vorrei ricordare al collega Manca e a tutta l'opposizione

Che dire poi di questo decreto milleproroghe, che insieme alla legge di bilancio e ancor prima al decreto aiuti-*quater* ci ha consentito di contrastare un quadro negativo molto pesante che c'era all'interno del nostro mercato nazionale? La riprova di ciò che sto dicendo la possiamo riscontrare attraverso le risposte positive che sono arrivate dai mercati, ma dobbiamo fare un'operazione verità, perché bisogna uscire dagli *slogan* e dalla retorica e inquadrare lo scenario

un'azione credibile per i mercati, che ha visto tutte le aste del debito pubblico superare la domanda rispetto all'offerta. Questo è qualcosa di importante perché sta a significare che i risparmiatori italiani si fidano dell'Italia e in particolare si fidano del loro Governo, che oggi li sta rappresentando in modo dignitoso. Parliamo di risparmi in un momento come questo, in cui non è facile avere la fiducia da parte dei contribuenti italiani. Parliamo dello *spread*: ricordate la drammatica estate del 2011, che ha visto cadere un Governo che era stato eletto legittimamente dal popolo italiano? Cosa si diceva fino a qualche mese fa? mercati, dello *spread*, dell'Europa e sembrava che questo Governo di destra-centro dovesse durare solo qualche settimana. Invece lo *spread* in questo momento testimonia lo stato di salute di ogni singola economia europea e anche del nostro Paese:

prospettive a quello che può essere il futuro della nostra Nazione. Potrei poi parlare della Borsa, che in appena cento giorni ha avuto volumi di scambi molto importanti, che superano di molto quelli legati al recente passato.

Ricordiamoci la montagna di risorse che abbiamo dato alle famiglie e alle imprese per sostenere una fase così delicata: 10 miliardi nel decreto-legge aiuti-*quater* e 20 miliardi nella legge di bilancio. Sto parlando di 30 miliardi che abbiamo destinato alle famiglie

grazie al Ministro e a tutti i commissari. Abbiamo raccolto i bisogni dell'Italia e abbiamo rispettato anche i tempi e questo non è un aspetto secondario, ma è di fondamentale importanza soprattutto perché rispetta la velocità che caratterizza i mercati finanziari nazionali.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ci tenevo molto, dopo questa giornata un po' faticosa, a svolgere questo intervento, perché credo sia giusto porre l'attenzione anche in quest'Aula su un caso che ha scosso la nostra comunità nel maggio del 2021. A cinque giorni dalla prima udienza del processo, trovo doveroso qui ricordare Saman Abbas. Saman è una ragazza pakistana di diciotto anni residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia,

Dietro la sua scomparsa sin da subito anche per gli investigatori ci sarebbe stato un movente assurdo: è stata uccisa dai familiari perché si sarebbe opposta alle nozze forzate con un cugino. Purtroppo, dopo mesi di ricerche e indagini, all'inizio di quest'anno abbiamo avuto la conferma di ciò che tutti temevamo: i resti umani ritrovati in un casolare di Novellara ci dicono che Saman è morta. Il processo chiarirà le responsabilità penali, ma gli elementi indiziari ci dicono che siamo di fronte a un caso assurdo, ad una morte ingiusta per ragioni altrettanto assurde. Saman è morta perché voleva essere una donna libera, perché aveva avuto il coraggio di denunciare all'età di diciassette anni i maltrattamenti in famiglia, l'induzione al matrimonio. Saman chiedeva di essere libera, di scegliere chi amare e chi non amare e io trovo sia importante ricordarla in quest'Aula, perché in Italia purtroppo sono tantissime le donne come Saman, vittime dell'indottrinamento religioso, vittime di una subcultura che non lascia libertà di scelta, donne invisibili, vite invisibili, sulle quali oggi con questo intervento vorrei che fosse fatta luce. Abbiamo un compito fondamentale: investire ora e sempre in cultura e in prevenzione. Mai più deve accadere che una donna, una qualsiasi persona sia obbligata e costretta a legarsi in una relazione imposta. Mai più deve deve accadere di morire per una ragione simile. Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di portare in quest'Aula questo caso e di far luce sulla storia di tante donne invisibili ai nostri occhi. Abbiamo un enorme lavoro da fare affinché sia fatta giustizia per Saman e per tante donne che come lei hanno il diritto di sentirsi libere di scegliere chi amare.